nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 495, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, interviene sulla materia dell'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese e ha la finalità di rafforzare la tutela del professionista. In particolare, il disegno di legge contiene la definizione di equo compenso, che è un compenso che dev'essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme a parametri per la sua determinazione.

professione. Per le professioni non ordinistiche, queste determinazioni sono previste da decreti del Ministero dello sviluppo economico. La disciplina si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che riguardano quindi prestazione d'opera intellettuale, che trovano fondamento in convenzioni e che siano svolte in favore di imprese bancarie o assicurative, nonché di imprese che l'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Viene estesa poi la disciplina dell'equo compenso anche alle prestazioni rese nei confronti della pubblica amministrazione, anche delle società a partecipazione pubblica. Nel dettaglio, il disegno di legge prevede la nullità di clausole che non prevedono compenso equo e proporzionato e viene elencata nella norma una serie di di pattuizioni. *In primis*, sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi previsti dai parametri. Si prevede poi la nullità di alcune pattuizioni

Si vedano, per esempio, le pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti o che impongono l'anticipazione di spese o che attribuiscono al committente o cliente vantaggi magari anche sproporzionati. Vi sono anche altri tipi di condotte,

del cliente di una somma in favore del professionista pari al doppio della differenza, quindi una sorta di indennità aggiuntiva.

modifica, per il cessare degli effetti dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2022 (la cosiddetta riforma Cartabia),

esprimere pareri, formulare proposte e segnalare pratiche elusive al Ministro della giustizia. L'articolo 11 è importante perché reca una disposizione transitoria in base alla quale queste norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore. La Commissione ha pertanto approvato il testo proveniente dalla Camera di deputati senza ulteriori modifiche, salvo questo ricordato riferimento normativo contenuto all'articolo 7.

lavoro autonomo e sulla possibilità anche per i professionisti di lavorare, pur nella libertà della loro professione, senza essere indotti, nel contesto di un mercato caratterizzato da una certa concorrenza,

intervengo in Aula in materia di equo compenso, giacché non è la prima occasione in cui il Parlamento si confronta su questo tema. Desidero fare mie le parole della Consulta sul lavoro autonomo e le professioni, indirizzate al Governo e al Parlamento in un documento nel quale si legge: «È urgente una regolazione dell'equo compenso delle prestazioni professionali, da lungo attesa. La disciplina attualmente vigente appare complessa, limitata sotto il profilo del campo di applicazione, oltre che inefficace per carenza di strumenti di controllo». Queste parole hanno trovato pieno ascolto e pieno riscontro nella proposta di legge che oggi sottoponiamo all'attenzione del Senato. Infatti, a quattordici anni di distanza dalle famose lenzuolate e a otto anni dall'abolizione delle tariffe, la liberalizzazione che avrebbe dovuto mettere

di sostenere la propria professione. Si badi bene: non è questa una battaglia sindacale, non è una battaglia di categoria. È una battaglia per la tutela effettiva dei diritti delle prestazioni professionali, perché - Presidente, mi permetto di dirlo con cognizione di causa, come tanti colleghi che in quest'Aula si sono occupati del provvedimento - sostenibilità della professione e qualità della prestazione sono due facce della stessa medaglia. Non ammetterlo è pura ipocrisia ed è ancora più ipocrita farlo in Italia - e sono certa che nessuna delle forze parlamentari rappresentate in quest'Aula lo farà dove la contrattazione collettiva copre oltre il 90 per cento dei lavoratori, rispettando a pieno la direttiva europea, mentre i professionisti lottano ogni giorno con contrattazioni al ribasso, con bandi di pubblica amministrazione che addirittura vorrebbero il lavoro gratis. Con questa legge daremo un taglio al doppiopesismo in danno ai lavoratori autonomi, tracciando un primo e importante perimetro di tutele.

È un provvedimento che già nella scorsa legislatura - lo ricordo, perché è una proposta di legge che gode di quella corsia preferenziale riconosciuta dal nostro Regolamento, poiché identica a un testo già approvato nella precedente legislatura - cominciò il suo *iter* in Aula grazie a una richiesta dell'allora capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida, che ne ottenne la calendarizzazione. Già nella XVIII legislatura, però, consapevoli dell'opportunità di fare di questa proposta di legge non una bandiera, ma piuttosto un testo sul quale lavorare tutti insieme, rinunciammo alle primogeniture condividemmo quello che era l'originario testo Meloni con tutte le forze politiche. L'importante era che ciascuno desse un contributo. Per questa ragione, il disegno di legge che oggi ci apprestiamo a votare è già il frutto di una sintesi, perché in questo testo ci sono emendamenti di tutte le forze politiche, che sono state approvati nella scorsa legislatura. Non c'è quindi la volontà di mettere bandierine sulle spalle dei lavoratori autonomi: lo abbiamo dimostrato quando eravamo l'unica forza di opposizione, lo faremo oggi che siamo la prima forza politica della Nazione e impediremo a chiunque altro di farlo. farlo. È importante ricordare che, rispetto alle iniziali previsioni, questo disegno di legge naturalmente si estende agli avvocati e ai professionisti iscritti a ordini e collegi, ma, grazie alla norma prevista nel comma 3 dell'articolo 1, anche alle professioni associate non regolamentate, di cui alla legge n. 4 del 2013. In Italia nessuno resta indietro. Le clausole di nullità, previste dall'articolo 3, sono uno strumento importantissimo, forse il cuore di questa proposta di legge, perché prevedono la possibilità di far valere la nullità di un contratto. Sono lo strumento messo nelle mani del contraente più debole, che è proprio colui che noi vogliamo tutelare. Lo abbiamo fatto senza cedere ad alcun tipo di pressione, confrontandoci con tutte le categorie coinvolte, e siamo consapevoli che questa proposta di legge rappresenti un punto di equilibrio pienamente soddisfacente per gli obiettivi che intende perseguire. Ne siamo talmente convinti, signor Presidente, che già nella scorsa legislatura accettammo di prevedere che vi fosse un osservatorio che coinvolge tutti; un osservatorio che, nella formulazione che abbiamo modificato nella scorsa legislatura, consentirà di verificare gli effetti applicativi di questa norma, che non resterà priva di controllo, perché la sua efficacia sarà vagliata e valutata, e naturalmente accompagnerà le riflessioni del legislatore. Infatti, non siamo infallibili e ne siamo consapevoli, ma piuttosto che rinunciare a fare qualcosa preferiamo dare un primo e importante segnale ai lavoratori autonomi, che aspettano da oltre un decennio. Di ciò siamo convinti e lo siamo ancora di più dopo l'esperienza che abbiamo vissuto durante la pandemia, quando i lavoratori autonomi furono destinatari di misure insufficienti, tardive e mai tempestive, che inevitabilmente hanno gettato centinaia di migliaia di partite IVA, con le loro famiglie, nella disperazione.

di tutte le associazioni, di tutte le categorie e di tutti gli organi istituzionali e associativi, per capire quale fosse la sintesi migliore, e riteniamo che la migliore sintesi possibile sia condensata nei 13 articoli di cui si compone il disegno Non è infatti un testo fatto di poche righe, ma al contrario contempla le più svariate esigenze, idonee a perseguire gli obiettivi che ci poniamo; il primo fra tutti è quello di evitare la proletarizzazione delle professioni, che a causa di una liberalizzazione sfociata in deregolamentazione affligge la nostra Nazione.

con la consapevolezza che questo disegno di legge costituisce una sintesi, che abbiamo condotto già nella scorsa legislatura con il vice ministro Sisto e con tanti altri colleghi, che in questi giorni hanno partecipato al dibattito in Commissione e in Aula. Desidero concludere ringraziando tutte le forze politiche per il voto unanime che daranno al disegno di legge in esame, targato Fratelli d'Italia e firmato da Giorgia Meloni. inoltre confermare a tutti ampia disponibilità al dialogo e al confronto, una volta che gli effetti applicativi di questa legge avranno visto la luce. Ci saranno altri momenti di confronto e ci sarà la possibilità di migliorare, ma qui e ora dobbiamo dare risposte a milioni di italiani.

Come già detto in sede di discussione dai nostri colleghi, avremmo certamente voluto che il testo venisse arricchito dei suggerimenti e degli apporti dell'avvocatura, dell'organismo congressuale forense, del movimento forense e degli stessi sindacati che tutelano il lavoro autonomo.

a ordini o collegi si fa riferimento a regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti dal Ministero vigilante sulla professione. Voteremo a favore perché, nonostante le lacune nell'ascolto e nella comprensione di altri autorevoli punti di vista in materia, riconosciamo al provvedimento il merito di voler tutelare alcuni settori del lavoro intellettuale, quando questo è svolto in convenzione con le imprese bancarie e assicurative e con le grandi imprese. non possiamo non sottolineare - come evidenzia ad esempio il punto di vista della CGIL del comparto - che tali migliorie si riferiscono solo ai rapporti di lavoro con grandi committenti e con le pubbliche amministrazioni, limitando nei fatti la platea dei lavoratori autonomi coperti. Inoltre, questo disegno di legge paradossalmente mette in difficoltà una parte dei lavoratori che dovrebbe tutelare, poiché attribuisce ai professionisti ordinisti una sanzione disciplinare in caso di accettazione di un compenso sotto soglia, pur essendo il professionista in posizione di debolezza rispetto al committente. Sarebbe stato necessario arrivare a una legge che potesse tutelare tutti i professionisti autonomi, soprattutto quelli contrattualmente più deboli. Il testo, per stessa ammissione del Vice Ministro intervenuto alla Camera dei deputati, si sarebbe certamente potuto migliorare, ma è stato lasciato così.

il Gruppo Per le Autonomie esprimerà un voto favorevole a un provvedimento che rappresenta un indiscutibile passo in avanti, perché restituisce dignità ai professionisti e ne valorizza il ruolo sociale, economico e istituzionale. Troppo spesso gli interventi sui lavoratori autonomi si concentrano sulla fascia alta, su quelli cioè che hanno già un'attività avviata e registrano un buon fatturato. È il caso, ad esempio, dell'estensione della *flat tax*, che ha portato un beneficio fiscale a coloro che annualmente fatturano più di 65.000 euro, ma il mondo delle libere professioni è fatto di persone che non raggiungono sempre certi *standard*, soprattutto negli anni iniziali della loro attività. Per questo il provvedimento che stiamo per votare introduce un principio fondamentale, soprattutto nei confronti dei giovani, che sono spesso i più sottoposti alle condizioni sfavorevoli del mercato. Il provvedimento infatti non si limita soltanto a definire un congruo valore delle prestazioni professionali, ma porta un equilibrio nelle situazioni in cui i committenti operano in una condizione di forza rispetto al professionista. In questi anni il rapporto dei lavoratori autonomi con la pubblica amministrazione è stato a dir poco tormentato: non solo la corsa al ribasso dei compensi, ma anche la lentezza e i ritardi nei pagamenti hanno fatto dello Stato italiano uno dei peggiori clienti. Alcuni ordini professionali hanno protestato più volte contro certi bandi che incitavano a una corsa al ribasso e sono riusciti in alcuni casi anche a tutelare i loro iscritti. Questo però, ovviamente, non è valso per tutti, perché ci sono ordini e categorie professionali meno forti e meno organizzati, per cui un intervento normativo che mettesse fine a questo *far west* non poteva più essere rimandato. Non vale neppure l'obiezione di alcuni, secondo i quali questo intervento è contrario al mercato e alla libera concorrenza, da un lato, perché non c'è libertà, laddove il rapporto negoziale è così sbilanciato nei confronti di una delle due parti, e, dell'altro, perché bisogna sempre tener conto della qualità della prestazione offerta, così come avviene nei bandi delle opere pubbliche, dove l'eccesso di ribasso è considerato la spia di una prestazione non adeguata dal punto di vista di materiali, sicurezza e tutela complessiva dei lavoratori. Il compenso adesso dovrà quindi essere calcolato incrociando qualità e quantità della prestazione offerta, pena la nullità di una pattuizione che violi questo principio. È chiaro che si tratta di un criterio non semplice da definire: ci sono sfumature e implicazioni e, non a caso, il dibattito nei due rami del Parlamento è stato ricco e articolato, ma quel che conta oggi è segnare un punto, quello per il quale se un professionista lavora molto, se è particolarmente competente o, ancora meglio, se soddisfa entrambi i criteri, deve avere un reddito adeguato alla sua preparazione e al suo impegno. Per tutte queste ragioni, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie sul provvedimento. Signor Presidente, con il nostro voto di oggi facciamo un altro passo avanti verso l'approvazione definitiva di una legge che può sembrare secondaria, ma non lo è affatto, ed è molto attesa da migliaia di liberi professionisti. Si tratta di un percorso iniziato molto tempo fa, nell'ottobre 2021, pertanto è una legge che rischiava di essere travolta, come spesso accade, dal cambio dal cambio di legislatura. Come Gruppo Azione-Italia Viva siamo stati da subito fra i primi sostenitori di questo provvedimento e siamo stati anche fra i primi Gruppi parlamentari a depositare disegni di legge che ricalcavano le norme già approvate dalla Camera. Questo perché riteniamo importante utilizzare una corsia preferenziale per arrivare presto all'approvazione del testo in esame, che restituisce dignità e potere contrattuale a una categoria - quella dei liberi professionisti - che è stata

le giuste ragioni di questo disegno di legge. Si tratta di un testo equilibrato, che intende difendere il lavoro dei liberi professionisti, il loro impegno, la qualità della loro opera nei confronti di committenti che in qualche modo, per il loro peso contrattuale, ottenere condizioni di svantaggio per la parte del professionista. Trovo che questo sia un qualcosa che ciascuno di noi, nel proprio quotidiano, ha potuto constatare come una pratica tutt'altro che secondaria. Qualcuno ha anche criticato questo disegno di legge. Si dirà che quello che stiamo facendo non è liberale, perché mettiamo in qualche modo un vincolo al mercato e alla libera contrattazione delle parti: non è così. Da liberale, difendo queste norme, perché appunto la contrattazione dev'essere realmente libera e, quando uno dei due contraenti ha una forza economica enormemente più grande di quella del professionista, è evidente che occorre un presidio che garantisca l'equità. È questo che abbiamo provato a fare, attraverso una legge la cui efficacia è stata circoscritta a un ambito d'applicazione preciso: le banche, le assicurazioni, le aziende con più di 50 lavoratori o con ricavi superiori ai 10 milioni di euro. Non si viola dunque in assoluto la libera contrattazione fra le parti, ma si prova ad improntarla a un principio di equità. La definizione del perimetro di imprese interessate a questa norma è assolutamente appropriata e poi, come sempre come sempre accade quando si approva una nuova legge, dovrà essere verificata e monitorata nella sua attuazione. Per questo abbiamo trovato ragionevole e ci siamo battuti per l'istituzione di un osservatorio nazionale presso il Ministero della giustizia: sarà questo l'organismo che, strada facendo, ci dirà i correttivi e ci suggerirà i miglioramenti da apportare alla legge. Condividiamo anche che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali siano aggiornati ogni due anni. Mi verrebbe da dire che si tratta che risponde al dinamismo del mercato. È molto opportuno aver espresso in maniera puntuale la nullità delle clausole vessatorie, come quelle che escludono il rimborso delle spese sostenute dal professionista o quelle che consentono al committente di modificare unilateralmente il contratto. Trovo importante aver ribadito che queste norme valgono anche quando il committente è la pubblica amministrazione. Sì, perché la pubblica amministrazione ha il dovere di dare il buon esempio e purtroppo - lo abbiamo visto anche nella prima fase di attuazione del PNRR - non mancano i casi nei quali è essa stessa invece a svilire e a non considerare il lavoro svolto dalle libere professioni. Questa legge s'inserisce nel solco di un'attività normativa che, soprattutto nelle ultime due legislature, ha cercato di inserire tutele che non erano previste per i lavoratori autonomi e i professionisti, allargando a questo mondo alcune tutele rilevanti. Penso al lavoro che è stato fatto sugli infortuni, sulla malattia, sulla maternità e sugli ammortizzatori sociali. È chiaro che tanto resta ancora da fare; nessuna legge è perfetta e tutto è perfettibile. Lo dico anche relativamente al dibattito che c'è stato su alcuni punti controversi alcuni punti controversi di questa legge, che sono stati oggetto di un'attività emendativa in Commissione. Penso, ad esempio, al tema delle sanzioni disciplinari per il professionista, al tema della non applicazione alle convenzioni in corso alla definizione del perimetro di applicazione della norma. Non su tutto abbiamo trovato una soluzione, proprio perché la scelta della maggioranza è stata quella di addivenire quanto prima a un'approvazione

non ha giovato; forse, se avessimo fatto un lavoro un po' più esaustivo, si sarebbe arrivati a un risultato di maggiore qualità, ma noi siamo abituati a prendere il lato positivo e a questo punto l'auspicio è che la Camera, che farà l'ultimo passaggio, licenzi al più presto questo provvedimento. Noi vogliamo il mercato, ma non vogliamo la giungla. È per questo che annuncio il voto favorevole di Azione-Italia Viva sul disegno di legge

Com'è stato detto da molti degli oratori che mi hanno preceduto stamane, il testo mira a rafforzare la tutela dei professionisti. Vari elementi insidiano in questa fase storica le professioni liberali, che sono invece un vanto della nostra storia, della nostra cultura e del nostro tessuto economico. Le professioni liberali sono una tradizione di secoli nel nostro Paese; risalgono addirittura al Medioevo le corporazioni, le gilde, che nel mio Veneto, al tempo della Repubblica di Venezia, si chiamavano però fraglie. Pensi, Presidente - mi piace sempre ricordarlo, quando parlo di questi temi nella mia città, Vicenza, lo statuto comunale prevedeva già nel 1264 otto fraglie, quelle dei mercanti, dei merciai, dei calzolai, dei macellai e degli albergatori, cui si aggiungevano i *collegia* dei giudici e dei notai. Dalla fraglia dei notai deriva oggi l'ordine degli avvocati, del quale ho l'onore e il piacere di far parte. *Lobby* economiche, grandi *corporation*, multinazionali e intelligenza artificiale mettono ora in discussione queste nostre tradizioni secolari sotto l'egida della *deregulation* senza regole e del mercatismo selvaggio. L'abolizione dei minimi tariffari ha esposto le professioni liberali a un'accettabile mortificazione, accettare contratti capestro, che ne sviliscono il ruolo e si pongono addirittura in contrasto con il principio implicito del nostro ordinamento, anche a livello costituzionale, secondo cui la prestazione professionale dev'essere retribuita in relazione alla qualità e quantità del suo valore economico. A questo fenomeno pone finalmente rimedio il testo in esame. Oggi c'è la possibilità di dare un forte segnale contro quella che in diverse occasioni - e ho sentito definirla così anche da altri oratori oggi intervenuti oggi intervenuti - ho voluto chiamare la proletarizzazione delle professioni, il tentativo di trasformare i liberi professionisti in parasubordinati. A questo tentativo ci opporremo con tutte le nostre energie: finalmente i contratti capestro non saranno più validi e non potranno più essere sottoscritti. La nostra speranza, signor Presidente, era quella di licenziare il testo senza modifiche e quindi approvarlo fin da oggi. Non è stato possibile, perché poi, nel corso dei lavori, si è ravvisata la necessità di una piccola modifica di coordinamento normativo, ma siamo fiduciosi che il testo, modificato solo con riguardo a questo dettaglio, troverà nell'altro ramo del Parlamento una scorciatoia per arrivare ad un'approvazione rapidissima. Certamente - e lo hanno ribadito anche altri oratori oggi intervenuti - il testo non risolve tutti i problemi delle categorie professionali, dobbiamo riconoscerlo:

e che in un futuro, spero prossimo, potremo definire in modo più compiuto. La prima riguarda la non retroattività della disciplina. Restano in vigore i contratti già stipulati, pure a condizioni capestro. Sarebbe stato opportuno probabilmente riuscire già in questo testo a sancire la nullità di quelle disposizioni. I contratti in essere sono evidentemente a tempo indeterminato e, se non vengono disdetti, manterranno efficacia a lungo. stabilito la retroattività della norma sull'equo compenso, credo che il bilancio dello Stato ne avrebbe tratto giovamento, perché le dichiarazioni Irpef dei professionisti nei prossimi anni sarebbero state sensibilmente superiori, con evidente beneficio anche per il gettito fiscale. Non è stato possibile: il Governo ci ha spiegato che ciò avrebbe comportato difficoltà insormontabili; ne prendiamo atto e lo accettiamo, ma ci impegniamo a ritornare sul punto alla prima occasione utile. Commissione, ma presumo anche in Aula, alcuni ordini del giorno, accolti dal Governo, che proprio a questo tendono. Il secondo punto oggetto di approfondimento in Commissione giustizia è la sanzione disciplinare, prevista per il professionista che comunque accetta clausole contrattuali vessatorie. Sul punto, in particolare il collega Bazoli ha molto insistito. Questa ipotesi sanzionatoria dev'essere però interpretata, almeno a nostro giudizio - e tengo a ribadirlo, affinché ne rimanga traccia nel Resoconto - non come una sorta di spada di Damocle che pende sul professionista, ma semmai come uno scudo, una tutela rafforzata che egli potrà invocare, per rifiutare, anche sul piano deontologico, contratti capestro che gli vengano imposti dal cliente. Peraltro, in condizioni particolari e provate, gli organi disciplinari degli ordini professionali potranno certamente lasciar andare esente da sanzione l'eventuale professionista che abbia agito in stato di necessità. In conclusione, signor Presidente, Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento tanto atteso dai professionisti di tutta Italia. Da sempre il nostro partito è vicino al ceto medio professionale e si batte per la sua tutela e la sua dignità.

per il puntiglio e la determinazione con cui ha seguito il testo, in questa, ma anche nella precedente legislatura. Una menzione speciale mi sento di farla anche alla relatrice, la senatrice Stefani, anch'ella avvocato, iscritta al prestigioso ordine di Vicenza, che ha guidato con competenza magistrale i nostri lavori in Commissione.

auguri al presidente Bongiorno, annuncio che il MoVimento 5 Stelle voterà favorevolmente al disegno di legge relativo all'equo compenso e non è difficile intuire il perché. Si tratta di un provvedimento molto sentito dalle categorie che vi vengono menzionate. Rappresenta un indubbio passo in avanti, circoscritto, ma essenziale, nei confronti di professionisti molto spesso sottopagati, soprattutto se giovani e agli inizi della carriera. meritevole di apprezzamento, in particolare laddove pone rimedio a situazioni di squilibrio che gravano nei rapporti contrattuali tra i professionisti e i cosiddetti clienti forti, quali banche e assicurazioni.

la maggioranza ha da sempre negato ogni possibilità di emendare il testo, in ragione della necessità di una sua pronta approvazione, onde evitarne il ritorno alla Camera per una seconda lettura. Per questa ragione, il MoVimento 5 Stelle ha richiesto in Commissione la sede deliberante, anche in virtù del fatto che sapevamo di essere gli unici ad aver presentato un emendamento che insisteva, nel merito, su un errore, figlio della sciatteria che, duole dirlo, sta contraddistinguendo la maggioranza relativamente alle tematiche della giustizia. *(Applausi)*. Consci del fatto che il testo sarebbe stato stato *obtorto collo* modificato, abbiamo richiesto il cambio di sede, solo al fine di velocizzarne l'*iter*. Governo e maggioranza da principio hanno negato tale possibilità, sulla base, tra l'altro, di un'invocata errata interpretazione della norma regolamentare, salvo poi assecondare un'ulteriore richiesta, che poi non è stata accolta dal Partito Democratico. Ora, in virtù dell'approvazione dell'emendamento a mia prima firma, il testo è stato modificato e pertanto vi sarà necessità di una lettura confermativa da parte dell'altro ramo del Parlamento. Mi chiedo, Presidente, una volta che il testo è stato aperto a modifiche, perché non sfruttare tale opportunità per migliorarlo definitivamente e consegnare ai professionisti una legge migliore ed effettivamente ineccepibile. Non è chiaro perché i colleghi della maggioranza si siano incaponiti nel non procedere alle modifiche che loro stessi avevano indicato negli ordini del giorno approvati in Commissione; o meglio, l'abbiamo capito molto bene: bene: non hanno proposto emendamenti, confidando nel fatto che il testo non sarebbe stato modificato e che quindi l'unico modo per migliorarlo sarebbe stato approvare gli emendamenti del MoVimento 5 Stelle. peraltro, andavano nella direzione dei temi trattati dai loro stessi ordini del giorno, ovvero eliminare le sanzioni ai professionisti che accettano compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai decreti e un'adeguata normativa transitoria. Se questo inciampo costituisse un *unicum*, non ci sarebbe da alzare polveroni, ma purtroppo - non so se dire per fortuna - ciò sta avvenendo con cadenza preoccupante: sono infatti fin troppe le questioni che ormai ci fanno pensare a una totale inettitudine da parte del Governo nelle materie afferenti la giustizia. L'omicidio nautico ve l'abbiamo riscritto, ci siamo poi accorti che non sapevate neanche copiare, infatti ci avete perfino copiato la brutta copia del neointrodotto delitto di *rave party.* Avreste fatto meglio a prendere in considerazione il nostro emendamento soppressivo, chiaramente prioritario rispetto a quello sostitutivo. Il disegno di legge governativo sul cambio di regime di procedibilità prende spunto dal disegno di legge a prima firma del senatore Scarpinato, depositato qui in Senato molto prima rispetto a quello governativo, e, visto che siete attenti a come lavora il MoVimento 5 Stelle relativamente alla giustizia, vi suggerisco di prendere spunto dalla nostra agenda politica e vi indico la strada da seguire: prima di tutto, adottare iniziative normative volte a superare l'istituto dell'improcedibilità, mantenendo ferma la disciplina della prescrizione dei reati come introdotta dalla legge spazzacorrotti; astenersi da qualsiasi intervento volto a riformare la disciplina delle intercettazioni, in modo da restringerne l'utilizzo o depotenziarne l'efficacia; adottare iniziative normative per modificare l'istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello, ripristinando le esclusioni dell'applicazione agli imputati per reati di particolare gravità; non intervenire sul delitto d'abuso d'ufficio e sul delitto di traffico di influenze e invece normare *lobby* e conflitto di interessi; assumere con la massima determinazione iniziative efficaci, volte al contrasto della violenza contro le donne, al fine di ridurre effettivamente il numero dei femminicidi riprendendo il percorso segnato dal codice rosso e proseguito dalla Commissione d'inchiesta sul femminicidio; rispettare integralmente, per quanto di competenza, il Titolo IV della Costituzione, laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura, nonché astenersi dal dare seguito a qualsivoglia proposta normativa di separazione delle carriere dei magistrati e di eliminazione mantenere e rafforzare gli strumenti di contrasto previsti dalla legislazione antimafia, in particolare salvaguardare il regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; in ultimo, tornare a investire nel comparto giustizia per rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadini quale unico vero antidoto alla lunghezza dei processi penali, colmando le scoperture e le vacanze degli uffici giudiziari attraverso una massiccia e e mirata attività assunzionale in continuità con le leggi di bilancio degli anni 2018 e 2020. Siamo certi, in tal modo, che il risultato sarà quantomeno soddisfacente. Stiamo approvando il disegno di legge relativo all'equo compenso. Vigiliamo tutti, a cominciare dal Ministero, affinché tali disposizioni siano concretamente applicate, anche perché bisogna sempre tenere gli occhi bene aperti. Abbiamo constatato che, proprio mentre si discute di equo compenso, il Ministero dell'università e della ricerca cerca 15 esperti di elevata specializzazione da inserire *full time* a costo zero: altro che equo compenso,

La dichiarazione di voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle l'ho fatta in premessa, perché avevo il timore che lungo il cammino avrei magari cambiato idea. *(Applausi)*.

rappresenta un indiscutibile passo in avanti per restituire dignità al professionista, valorizzandone al contempo il ruolo sociale, economico e istituzionale,

ottenuta - si badi - senza il ricorso a mobilitazioni di piazza, scioperi o picchetti, perché la categoria che in questo caso ci interessa è quella dei professionisti. Tuttavia, le similitudini con altre categorie di lavoratori riguardano sempre la presenza nel rapporto contrattuale di un contraente forte, il quale il più delle volte, nella fase dell'affidamento dell'incarico, è capace di imporre onorari e clausole standardizzati e condizioni del tutto indignitose, che riguardano ampi strati delle giovani leve professionali, che sono incapaci di rifiutare l'opportunità offerta, perché già alle prese con la difficile quadratura del proprio bilancio reddituale. il voto odierno, infatti, si determina un successo sul terreno del recepimento legislativo delle istanze provenienti dal mondo del lavoro professionale e dalle sue rappresentanze. Dal tempo delle grandi mobilitazioni e delle conquiste normative e salariali non assistevamo alla traduzione in legge di diritti e previsioni così incisivi afferenti a un vasto strato del mondo lavorativo. Per dimostrare ciò che affermo, bastino soltanto le parole utilizzate da alcuni rappresentanti delle categorie professionali. Ad esempio, per il mondo dell'avvocatura si parla non soltanto del

Per quanto riguarda i geometri, si parla invece di un vero e proprio spartiacque, che riallinea correttamente il principio dell'equo compenso al mercato e alla concorrenza. Inoltre, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, che rappresenta come questa sia una tappa importante sulla via di un più ampio riconoscimento di tutele per i professionisti, la definisce un'inversione di tendenza molto significativa nell'atteggiamento della politica nei confronti dell'universo delle libere professioni. Potrei continuare con gli ingegneri, i quali parlano di un indiscutibile passo in avanti, che non solo restituisce dignità al professionista valorizzandone il ruolo sociale, ma rafforza anche quello economico e istituzionale e difende il diritto dei cittadini a ricevere servizi di qualità. Effettivamente, dopo l'importante novità della cosiddetta tassa piatta o *flat tax,* questa normativa appare la seconda più importante misura a sostegno dell'ottimizzazione della redditività delle attività professionali. se i parametri rappresentano importi e quantificazioni stabiliti per ogni categoria e attività attraverso un decreto ministeriale,

Il disegno di legge sull'equo compenso è stato approvato dalla Camera dei deputati e nel suo attuale *iter* in sede redigente come tutti i movimenti e i partiti qui rappresentati premano affinché si abbia un veloce via libera. Ovviamente stona, purtroppo, la circostanza che all'interno del testo una norma, abrogata nel convulso succedersi di riferimenti normativi, abbia aperto la strada all'odierna necessità, peraltro tempestiva, di una modifica che impone un nuovo passaggio un nuovo passaggio parlamentare, ossia il ritorno in terza lettura alla Camera. Ho ascoltato alcune delle osservazioni fatte dai colleghi prima di me e vorrei dire che sì, è vero, molto si poteva ancora fare, ma devo dire che in Commissione giustizia il vice ministro Paolo Sisto, come ricordava poc'anzi il collega Zanettin, ha anzitutto rassicurato - e ne è testimonianza l'approvazione di ben tre ordini del giorno presentati dalla Lega

all'eliminazione della previsione che impone agli ordini e ai collegi professionali di adottare sanzioni disciplinari, perché questo stride evidentemente con la mancata possibilità di fare altrettanto per le professioni non regolamentate da riferimenti ordinistici; all'allargamento della norma a realtà di committenti oggi escluse; ed ancora, a un ordine del giorno che ha inteso individuare l'attenzione del Governo sulla possibilità di ampliare con altre rappresentanze i componenti dell'Osservatorio introdotto dalla legge. È dunque l'occasione sin d'ora per lanciare altre sfide in favore delle professioni, le quali trovano ancora oggi nelle norme e nei codici dello Stato relitti residui che non hanno più motivo di esistere e che appaiono solo come una rispettosa tolleranza della tradizione dottrinaria. Faccio solo riferimento, ad esempio, al caso delle prescrizioni presuntive, che sono superabili addirittura con il deferimento di un giuramento decisorio, cioè un relitto del passato che oggettivamente, per quanto attiene alle professioni, forse oggi potremmo anche decidere di ripensare. Concludo con i ringraziamenti alla relatrice, la mia collega Erika Stefani, e non posso ovviamente non fare riferimento al bellissimo regalo che quest'oggi porterà a casa la collega, presidente Giulia Bongiorno, per il giorno del suo compleanno, in occasione del quale le rivolgo anch'io gli auguri del Gruppo Lega. sempre al fianco delle partite IVA esercenti attività professionali, e non solo, e naturalmente di quelle le ordinistiche e non, crogiuolo di grandi e complessi saperi. Signor Presidente, anche il Partito Democratico, come gli altri Gruppi parlamentari, voterà a favore di questo testo di legge, anche se non siamo molto soddisfatti di come si è arrivati in Aula. Voteremo a favore intanto perché condividiamo gli obiettivi di questo disegno disegno di legge, ossia garantire e riconoscere ai professionisti un compenso dignitoso, tenuto conto del fatto che, dopo che furono abolite le tariffe minime e massime negli anni scorsi a seguito dell'approvazione di norme che tutelavano il mercato e andavano nella direzione voluta dalle regole dell'Unione europea, troppo spesso committenti forti hanno imposto condizioni contrattuali ai professionisti che sono anche andate a ledere la dignità del lavoro dei liberi professionisti. Condividiamo l'obiettivo di garantire invece compensi adeguati e proporzionati alla dignità del lavoro fatto dai liberi professionisti e devo dire che ci piacerebbe che lo stesso zelo che ha messo la maggioranza in questo disegno di legge ci fosse anche per tutelare i salari dei lavoratori dipendenti *(Applausi)*, perché su questo ci pare invece che ci sia una distrazione che francamente non comprendiamo.

che migliorare, sistematizzare ed estendere i principi che furono già introdotti nell'ordinamento italiano dalla legge Orlando due legislature fa. L'equo compenso c'è già nel nostro ordinamento. Questo disegno di legge - ed è una cosa positiva - migliora l'impianto introdotto nell'ordinamento della legge Orlando. Non si tratta di una rivoluzione, ma del miglioramento di qualcosa che facemmo già noi due legislature fa. Questo credo sia opportuno ricordarlo. Dicevo però che, per quanto condividiamo sia gli obiettivi sia l'impianto di questa riforma, che appunto migliora quello della legge Orlando, non siamo particolarmente soddisfatti di come ci si è arrivati, perché riteniamo che il che il testo fosse migliorabile in alcuni dettagli significativi. Per questo avevamo proposto alcuni emendamenti in Commissione,

alcuni ordini del giorno che richiamavano il contenuto di quegli emendamenti e sui quali lo stesso Governo ha dato parere favorevole. Allora, come mai non sono stati approvati questi emendamenti? Ci è stato spiegato dalla maggioranza e dal Governo

senza modifiche, perché eravamo alla fine della legislatura e non c'era più tempo, ora siamo all'inizio della legislatura e c'è tutto il tempo che si vuole per migliorare un testo, se si ritiene che sia migliorabile. Non si capisce quindi perché su questo testo in particolare

venir meno questa giustificazione che noi stessi non condividevamo. È successo che nel testo che è stato portato qua c'era un baco,

non ci è stato consentito di fare queste modifiche su temi sui quali la stessa maggioranza ha presentato ordini del giorno, sui quali il Governo ha espresso parere favorevole. Perché non ci è stato consentito di fare quelle due o tre modifiche sulle quali c'era l'accordo di tutti, tenuto conto del fatto che il testo tornerà comunque alla Camera? La risposta è «boh». Non lo sappiamo e non abbiamo capito la ragione per cui ci è stato impedito di migliorare un testo che, per carità, è un grande passo in avanti rispetto alla situazione attuale (quindi noi lo voteremo), ma che inevitabilmente dovrà essere sottoposto a ulteriori correzioni con altri interventi legislativi. Perché? Che modo di legiferare è questo? Per un semplice puntiglio non si sono approvate modifiche sulle quali le stesse categorie professionali ci avevano chiesto di intervenire. alla sanzione disciplinare per i professionisti che sottoscrivono un accordo che vìola i principi dell'equo compenso, mi ricordo la *ratio* che aveva giustificato questo inserimento. Era quella di dare ai professionisti uno scudo

Se per caso però un professionista, obbligato dallo stato di necessità, firma comunque un accordo che viola l'equo compenso, a quel punto è fregato, perché non potrà più denunciare la convenzione che viola l'equo compenso, altrimenti sarà sottoposto a sanzione disciplinare. Capite che è una contraddizione, un errore, un altro baco di questa legge? Infatti,

fondamentale di civiltà rispetto al lavoro dei liberi professionisti, che aveva subito uno, due, forse tre passi di più), nel momento in cui l'Italia aveva pensato che, con la liberalizzazione delle tariffe, i liberi professionisti sarebbero stati proprietari del loro destino, applicando quelle che meglio rappresentassero il loro lavoro, nei confronti dei committenti, pubblici o privati che fossero. fossero. Abbiamo visto invece come negli ultimi vent'anni i liberi professionisti, che nel secolo scorso erano la parte forte, quando sottoscrivevano un contratto con l'altra parte che li incaricava di qualcosa, sono diventati la parte debole, anzi debolissima, anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il lavoro dei liberi professionisti non può essere valutato a seconda di quanto poco fanno pagare a seconda di quanto poco le loro prestazioni vengono contabilizzate da un ente, una grossa assicurazione o una banca. Capita spesso che i liberi professionisti, obbligati a sottoscrivere

conseguente prestazione economica, che dev'essere congrua rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Ad esempio, nei confronti della pubblica amministrazione, sulla base minima prevista dall'equo compenso, renderà tutti uguali e le pubbliche amministrazioni saranno libere di scegliere i liberi professionisti non solo in funzione di quanto meno fanno pagare, ma, data la base minima, considerando la loro bravura e il rapporto di fiducia che hanno con la pubblica amministrazione. Questo succederà anche con le banche e con le assicurazioni. È quindi un fondamentale passo avanti per il rapporto tra liberi professionisti, pubbliche amministrazioni e aziende molto solide.

anni lavorerà per capire come la legge è stata applicata e quali misure sia necessario porre in essere per modificarla e renderla così ancora migliore.

dei liberi professionisti? Ebbene, penso che questa legge sia, sì, migliorabile (lo pensiamo tutti e lo abbiamo anche detto), ma credo sia molto più importante approvarla in tempi molto brevi per far sì che la vita e il rapporto tra i liberi professionisti e chi dà loro gli incarichi, compresa la pubblica amministrazione, cambino radicalmente. Questa è una rivoluzione copernicana per quanto riguarda i liberi professionisti, di cui anch'io faccio parte, e devo dirmi molto soddisfatto che questo provvedimento venga approvato, perché non saremo più costretti a

magari, accetterebbe tariffe non corrispondenti all'equo compenso solo per ottenere l'incarico. Possiamo migliorare su questo aspetto? Penso di sì. Penso anche che questa mattina, in questa sede, dove tutte le parti politiche che compongono il Senato si sono dichiarate favorevoli - con qualche distinguo su cosa si potesse fare di più o di meno - non maggioranza e Governo di sciatteria. Dispiace, perché parlare di sciatteria è un'offesa e, per come sono andati i lavori in Commissione giustizia e per come sono andati ancor prima, abbiamo riconosciuto che, per la normativa che è stata approvata successivamente, quell'articolo aveva bisogno di essere modificato; non siamo caduti dal melo e non abbiamo aperto la bocca tanto per dire che non ce n'eravamo accorti. Essere accusati di sciatteria denota l'astio di chi forse vorrebbe essere al nostro posto ed è stato condannato dagli italiani a non esserci più. Respingiamo anche la vostra proposta di stare alla vostra agenda sul campo della giustizia, perché abbiamo un Primo Ministro, un Ministro,

Con questo voto unanime del Senato, risulta assorbito il disegno di legge n. 182.

di legge n. 495. DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista

la ratifica dell'accordo in questione si colloca nell'ambito di un processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam. L'accordo inoltre è finalizzato a consentire un miglioramento del contesto entro cui si collocano gli investimenti europei in Vietnam, assicurando agli investitori europei una condizione di non discriminazione rispetto agli investitori locali e fissando una serie di tutele a loro vantaggio, a partire da quelle in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. Il testo offre altresì agli investitori la possibilità di ricorrere a un vero e proprio sistema giurisdizionale di tutela degli investimenti, incentrato su un apposito tribunale permanente. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Signor Presidente, devo dire di essere particolarmente lieto di poter intervenire su questo disegno di legge di ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti in Vietnam,

è uno dei principali esportatori al mondo, collocandosi tra l'ottavo e il nono posto. Possiamo dire dunque che la nostra economia si regga sostanzialmente sull'interscambio estero: se andiamo a guardare la nostra bilancia commerciale

vendendo all'estero più di quanto compravamo, sono state la ragione per la quale siamo riusciti ad attraversare le varie crisi economiche che si sono susseguite dall'inizio di questo millennio. In questo modo, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a venirne fuori in qualche maniera. Eppure gli accordi di libero scambio, che per loro definizione servono ad aiutare le nostre imprese a vendere i nostri prodotti nel mondo e servono a rendere la vita più facile agli imprenditori che vendono la nostra moda, il nostro agroalimentare, la nostra meccanica e la nostra farmaceutica, farmaceutica, sono stati la principale o una delle principali vittime della canea populista che si è impadronita di questo Paese e del mondo negli ultimi anni.

anche a stabilire legami politici. Come diceva infatti il filosofo francese Frédéric Bastiat nell'Ottocento, dove non passano le merci passano gli eserciti e mai come in questo momento dovremmo ricordarcene. la ragione per la quale un accordo di libero scambio è fatto da una parte che serve alla promozione del commercio internazionale e da un'altra che serve alla protezione degli investimenti, perché è chiaro nessun investitore andrebbe a investire all'estero, dovendo poi in caso di controversia andare a difendersi davanti a un tribunale del Paese ospite. È una situazione del tutto sbilanciata e quindi evidentemente gli accordi di libero scambio devono prevedere una parte in cui si dica che, se l'investitore va in un certo Paese e c'è una controversia, quell'investitore va protetto e noi,

ascoltano i suggerimenti provenienti dall'economia e dagli esperti, l'accordo con il Vietnam contiene una significativa novità, che vorrei segnalare a tutti i colleghi. Questo è uno dei primi accordi stipulati dall'Unione europea nei quali è stato superato il vecchio sistema ISDS (che sta per *Investor-State

protette anche lì. Per capirci, prima del CETA, il prosciutto di Parma in Canada si vendeva come *original prosciutto*, perché il marchio Parma era stato registrato da un'azienda canadese. Ebbene, nonostante tutto dica che questo è un buon accordo, noi ancora non riusciamo a ratificare la parte

quando noi italiani, invece di negoziare da soli gli accordi di libero scambio, possiamo sederci al tavolo col peso di 500 milioni di abitanti e consumatori dell'Unione europea e offrire sbocco vero un mercato così importante, le condizioni che spuntiamo sugli accordi di libero scambio sono ovviamente molto migliori

Di questo Governo sapevamo che avrebbe fatto il blocco navale, che avrebbe bloccato le accise e avrebbe fatto tutta una serie di misure che non abbiamo visto. Questo sarà chiaramente l'ennesimo cambio di idea del Governo Meloni, ma, quando

di cui nessuno si è mai lamentato, forse perché non c'era polemica politica da fare in queste Aule. Ci si ricorda infatti di essere *no global* e contro il libero commercio soltanto quando c'è da fare polemica politica; quando entra in vigore un accordo con il Giappone, che non deve passare per le Aule del Parlamento, nessuno dice niente. dice niente. Noi naturalmente voteremo a favore di questa ratifica. Lasciatemi infine dire: proteggiamo il nostro commercio internazionale. Via le ideologie, via il populismo. Le misure che fanno bene al Paese siano approvate con la più larga più larga maggioranza possibile.

parte, aspetti preminentemente tecnici dei rapporti che l'Unione europea e i suoi Stati membri intrattengono con Paesi terzi e, dall'altra, l'adesione a convenzioni internazionali su specifiche tematiche. Sarebbe sbagliato però non cogliere anche la portata tutta politica di alcune di queste ratifiche, soprattutto perché due di esse riguardano accordi sulla protezione degli investimenti sviluppati con realtà asiatiche strategiche quali la Repubblica di Singapore e la Repubblica socialista del Vietnam. Questi due accordi non solo assicurano un elevato grado di tutela per gli investimenti, garantendo agli investitori europei, e quindi italiani, un trattamento non discriminatorio, ma rappresentano una proiezione geoeconomica dell'Europa e delle sue realtà in un quadrante dello scacchiere mondiale assai importante e significativo.

accordi in questione assumono quindi una notevole rilevanza per molteplici ragioni. In primo luogo, si inseriscono in un contesto di intense relazioni economico-commerciali già in essere tra l'Unione europea e il gruppo dei Paesi del Sud-Est asiatico, l'Association of South-East Tanto il Vietnam quanto Singapore rappresentano il principale *partner* dell'Unione. Hanoi conosce una crescita significativa e un aumento degli investimenti diretti esteri con un crescente interscambio proprio con l'Italia. Singapore, realtà esportatrice per ben 8.000 imprese italiane, riveste un evidente ruolo strategico non solo per il proprio mercato locale, ma anche - e aggiungo soprattutto - come porta d'accesso al più vasto mercato del Sud-Est asiatico in ragione dell'altissimo livello qualitativo che caratterizza le sue infrastrutture e i suoi apparati logistici. È quindi evidente, da questi numeri del complessivo quadro geoeconomico e geocommerciale, che tali accordi non solo erano utili, ma necessari. Come sappiamo, le Nazioni asiatiche dipendono per larga parte dalla Cina per il loro commercio. Eppure, nonostante ciò, non intendono legarsi a questa sul piano geopolitico. Ecco perché, in secondo luogo, tali accordi hanno la rilevanza politica che richiamavo in premessa, perché interessano il rapporto con due realtà che vogliono coltivare a tutto tondo un rapporto privilegiato con l'Occidente e con l'Europa e che molto spesso - pensiamo a Singapore coltivano strette relazioni anche in funzione della loro strategia di difesa, specialmente per quanto concerne lo sviluppo della deterrenza militare. Le altre due ratifiche su cui il Senato è chiamato a pronunciarsi riguardano aspetti su cui, con tutta evidenza, non può che esserci comune sentire dell'Assemblea e di tutte le forze politiche. Tanto il tema della registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali regolati della Convenzione di Ginevra quanto la ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping* di Varsavia hanno al centro, seppur da punti di vista e prospettive diversi, la tutela della persona e del cittadino. Appare a noi tutti evidente che estendere il sistema di protezione a nuovi membri, omogeneizzare le legislazioni nazionali, snellire il sistema di registrazione e istituire un collegamento tra il sistema di registrazione La ratifica del protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Varsavia contro il *doping*, poi, è un dovere morale non solo per sanzionare una condotta illecita, contraria alla ragione ancor prima che al diritto e alla stessa idea di sport, ma soprattutto per tutelare la salute degli atleti di tutto il mondo. Annuncio così i quattro voti favorevoli del Gruppo Forza Italia.

un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie che tutela gli investimenti e pone gli investitori in una situazione di non discriminazione. Per tale ragione, annuncio il voto favorevole del Gruppo sulla ratifica

di nuove sostanze ritenute dopanti. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

ci sono stati più passaggi e più occasioni di approfondimento. In particolare, esse riguardano la protezione degli investimenti, la prima per quanto riguarda il Vietnam e la seconda per quanto riguarda Singapore, e sono state stipulate nell'ambito della politica commerciale, quindi, essendo comunitarie, dall'Unione europea e dagli Stati membri; essendo tipici accordi misti, hanno bisogno della doppia ratifica, quindi anche di quella dei singoli Parlamenti nazionali.

la legislazione italiana si ispira. Per dare completezza si arriva ad approvare anche la ratifica: è quasi un atto dovuto, così come la ratifica dell'Atto di Ginevra che, diversamente dagli altri due ambiti, cioè il Consiglio d'Europa

voto favorevole. Le due ratifiche in esame riguardano due Nazioni sicuramente importanti e molto diverse tra loro: da un lato, la Repubblica socialista del Vietnam e, dall'altro, Singapore, un po' l'alfa e l'omega di quel territorio, da un punto di vista economico e della loro della loro organizzazione interna. È chiaro che la protezione degli investitori e la creazione di tribunali terzi per le eventuali controversie che i nostri

che francamente non so da dove possa provenire, il racconto di un centrodestra e di una destra italiana che è molto lontano dalla realtà e dalla coerenza che ci ha sempre contraddistinto in tutti i campi,

Parlamenti nazionali. In questo quadro, ribadisco il voto favorevole su entrambi i citati provvedimenti da parte del Gruppo Fratelli d'Italia.

alla protezione degli investimenti, è esattamente identico, anche se non riguarda Singapore o il Vietnam, alla parte mancante del CETA. La parte sul libero scambio del CETA è già in vigore da cinque anni in esecuzione provvisoria, mentre manca quella sugli investimenti. Non capisco allora perché il Governo calendarizzi e porti in Aula la protezione degli investimenti con Vietnam e Singapore e non ci consenta di approvare quel pezzettino del CETA che ancora manca. Siamo soltanto undici Paesi: dato che avete fatto un'apertura, mi aspetto - lo dico alla Sottosegretaria - che il CETA finalmente arrivi in Aula molto presto. Dopodiché, per il suo tramite, Presidente, dato che il collega di Fratelli d'Italia che ha parlato prima di me ha detto che loro, sui trattati di libero scambio, sono stati sempre

*tweet* del 15 febbraio del 2017, alle ore 13,15, a firma di una tale Giorgia Meloni (non so se la conoscete, mi dicono che sia il Presidente del Consiglio dei ministri), che dice che il CETA, il trattato di libero scambio tra Unione europea e Canada,

anche in caso di giovane età, i ricordi possano sfumare, soprattutto quando sono sgraditi o quando si è fatto qualcosa che oggettivamente era contrario agli interessi nazionali, essendo noi un grande Paese esportatore, dire che un trattato di libero scambio

premi, come altri ciclisti hanno fatto in passato, ma che ha deciso invece di essere pulito fino alla fine, magari con una carriera sportiva più faticosa, ma più bella.

un'osservazione sul fatto che stiamo per approvare un Protocollo aggiuntivo che è datato 2004.

sta facendo atti di governo importanti. Voglio citare ad esempio una testimonianza concreta, avvenuta in questi mesi, ovvero l'accelerazione che il Governo ha imposto per l'approvazione del Piano nazionale delle malattie rare, che era scaduto nel 2016. Oggi votiamo quindi con molto piacere

oggetto e mi fa piacere che quello odierno non sia solo un atto formale. Dato che c'è la sensibilità da parte di tutti i colleghi di trattare questo argomento, mi piace ricordare che lo sport è soprattutto modelli etici da perseguire, rispetto dei valori,

Soprattutto sono da combattere la mentalità e la cultura, specie in quegli ambienti lontani dalle luci della ribalta e dalle competizioni internazionali, negli sport cosiddetti minori e amatoriali che spesso inducono gli atleti, anche inconsapevolmente, ad assumere sostanze che li portano a una vittoria con frode, quindi condotta sleale, ma anche nociva per la propria salute. Per questo, non solo formalmente, oggi, ma anche per il merito del tema, stigmatizzando

Grazie a tutti

Parto con una citazione di Edison: il valore di un'idea sta nel metterla in pratica. Questa non è una ratifica banale, ma molto importante: d'ora in poi sarà infatti più semplice la registrazione internazionale con un'unica domanda di disegni e modelli industriali. L'Accordo dell'Aja riguarda la registrazione internazionale e permette al titolare di un disegno o di un modello industriale di ottenerne la protezione in tutti i Paesi scelti tra quelli aderenti mediante un'unica domanda presso un solo ufficio, redatta in una sola lingua, pagando una sola volta le tasse in una moneta, il franco svizzero, salvo che la protezione non sia rifiutata dall'ufficio competente del Paese designato. Per renderlo possibile, il disegno di legge di ratifica modifica il codice di proprietà industriale. Le finalità principali di questo atto, che consta di 31 articoli strutturati in quattro capitoli, sono estendere il sistema delineato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri e mantenere la semplicità e la semplificazione del sistema. La previsione che le organizzazioni intergovernative possano aderire consente anche di creare un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i vari sistemi regionali. Le modifiche riguardano soprattutto l'articolo 3,

o un'effettiva organizzazione in Italia possano depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'ufficio internazionale oppure presso l'ufficio italiano brevetti e marchi. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati nell'Accordo del 1999. L'articolo 4 disciplina poi la durata della protezione dei disegni e dei modelli; in particolare, la protezione internazionale del disegno e del modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata conformemente alla durata massima della protezione. In sintesi, gli obiettivi principali di quest'atto consistono nell'estensione del sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri, in modo da facilitare l'adesione degli Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. Si è voluto naturalmente semplificare il sistema ed è stato consentito il collegamento di tutti i sistemi internazionali e regionali. Sulla questione però che mi sta più a cuore, con i colleghi del nostro Gruppo, abbiamo presentato un ordine del giorno, chiedendo al Governo di valutare anche l'adozione di ulteriori interventi che possano incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti. A tal proposito, ricordo che negli ultimi anni si è registrato un aumento delle domande di brevetti presentati dall'Italia. Il contributo maggiore è quello delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimiche e farmaceutiche. Dal punto di vista territoriale, la Lombardia è la Regione in cui si concentra la capacità innovativa più alta, seguita dall'Emilia-Romagna, dal Veneto, dal Piemonte e dalle altre Regioni. Da qui si evidenzia come vi siano grandi potenzialità nel nostro Paese e nel sistema Italia ancora da sviluppare su tutto il territorio nazionale. Nonostante i grandi sforzi, negli ultimi anni nelle classifiche che registrano la produzione di brevetti l'Italia è appena dietro rispetto ad altri Paesi industrializzati, come la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, la Cina. Questo comporta rischi per le nostre aziende che operano in un mercato sempre più globalizzato. Le principali analisi rilevano come aziende ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale abbiano maggiore capacità di creare sviluppo e ricchezza. Inoltre, il possesso di un buon portafoglio di brevetti è percepito dal mercato internazionale come la dimostrazione dell'alto livello di specializzazione e capacità tecnologica dell'azienda. Fondamentale è quindi l'adozione di misure e norme che facilitino e incentivino l'attività di ricerca delle imprese, per aumentare la capacità del nostro Paese di produrre nuovi brevetti, rendendo così il nostro sistema produttivo più competitivo sui mercati internazionali. Ringrazio naturalmente il Governo, che ha accolto quest'ordine del giorno. Non sprechiamo più tempo. Naturalmente, annuncio il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione su tutte le ratifiche all'ordine del giorno di quest'Assemblea.

Grazie a tutti

Onorevoli senatori, il 20 dicembre 2022, la Commissione affari esteri e difesa del Senato ha approvato all'unanimità una una risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta che hanno fatto seguito alla morte di Mahsa Jina Amini, una giovane iraniana di origini curde, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla cosiddetta polizia morale della Repubblica islamica, con l'accusa di aver indossato il velo in modo inappropriato. La morte della ventiduenne, sopraggiunta pochi giorni dopo, a causa delle violenze cui è stata sottoposta mentre si trovava in stato di fermo, ha dato il via a numerose manifestazioni pacifiche di protesta, che in breve tempo hanno assunto un'autentica dimensione di massa, interessando almeno 150 città e 140 università in ciascuna delle 31 province dell'Iran, dove hanno giocato un ruolo attivo non solo le donne, ma i cittadini espressione di tutti gli strati sociali. Piuttosto che aprirsi al mondo, il regime di Teheran ha deciso di usare il pugno di ferro. Ha scelto di sparare contro la sua gente e di dar corso a una rappresaglia che non ha scoraggiato e non sta scoraggiando nessuno, ma che, anzi, ha delegittimato ancora di più l'intero sistema teocratico, che soffoca le libertà personali e i diritti civili. Sin da subito, la Commissione affari esteri e difesa che ho l'onore di presiedere ha seguito con attenzione preoccupata l'evolversi degli eventi. Nel dicembre scorso abbiamo audito un gruppo di studenti iraniani che vivono in Italia. A quei ragazzi e a quelle ragazze, impauriti e al contempo orgogliosi, abbiamo manifestato tutta la solidarietà e la vicinanza, concordando sul fatto che la comunità internazionale, dopo aver espresso sentimenti di condanna, dovesse intensificare la pressione politico-diplomatica per fermare la spirale della violenza. Dai loro discorsi e dalle loro testimonianze ho tratto conferma che la brutalità e le intimidazioni non fermeranno l'anelito di libertà che muove il popolo iraniano. Il vento della storia sta soffiando forte in quel Paese ed è destinato a spazzare via l'illusione che tutto potrà continuare come se nulla fosse accaduto. Oggi prendo la parola in Aula nella certezza che le speranze di quei giovani non debbano essere deluse e che quei ragazzi non possano essere abbandonati e traditi. Sentimenti di forte inquietudine ho altresì espresso al Presidente della Commissione per la sicurezza e la politica estera dell'Assemblea consultiva della Repubblica islamica dell'Iran, nel rispondere alla lettera con la quale auspicava il rafforzamento delle relazioni bilaterali, anche attraverso l'utilizzo della leva della diplomazia parlamentare. Dal giorno della morte di *Mahsa Amini*, oltre 500 civili sono stati uccisi e almeno 20.000 giovani sono finite nelle famigerate carceri iraniane, dove - secondo le testimonianze - subiscono violenze brutali e a volte perdono la vita. Un sistema che uccide i suoi figli è eticamente e tecnicamente illegittimo. Un regime che colpisce e odia le proprie donne è anche antropologicamente innaturale. è molto probabile che quello stesso regime si stia avviando al limite della resistenza. Questa percezione viene corroborata dal fatto che, nell'utilizzo di ogni strumento per fermare le rivolte di popolo, in genere si usano i mezzi più oppressivi quando ogni altra forma di controllo risulta inefficace. È ormai certo, inoltre, che la battaglia contro il sistema sclerotizzato degli *ayatollah* non si combatta più solo nelle strade, dalla capitale al più piccolo dei luoghi periferici, ma che sia penetrata nelle menti e nei cuori e che si manifesti attraverso gesti eclatanti in ogni sede, anche fuori dai confini nazionali. È vivo il ricordo dei giocatori della nazionale di calcio iraniana che, ai Mondiali in Qatar, restano in silenzio e non cantano l'inno in segno di solidarietà ai manifestanti uccisi. Trasudano coraggio e dissenso nei confronti del regime i comportamenti della scalatrice Elnaz Rekabi e della campionessa di scacchi Sarasadat Khademolsharieh, che hanno gareggiato senza velo, a capo scoperto. Onorevoli senatori, il provvedimento giunto oggi all'esame dell'Assemblea impegna il Governo italiano a fare pressione su Teheran direttamente nelle sedi multilaterali

Occorre adoperarsi con la massima sollecitudine per scongiurare il rischio reale di nuove esecuzioni capitali. Servono iniziative e pressioni da articolare di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea e del mondo occidentale per indurre le autorità iraniane a garantire il pieno rispetto dei diritti umani verso i propri cittadini e verso le minoranze presenti nel Paese. È quanto ad oggi possiamo realisticamente fare: schierare le istituzioni democratiche, parlamentari e rappresentative senza equivoci dalla parte del popolo iraniano. Il nostro è solo un primo passo possibile, il tassello di un mosaico più ampio che dev'essere composto, un mosaico di solidarietà, vicinanza e sostegno concreto a chi rischia la propria vita in nome della libertà.

desidero ringraziare il presidente della Commissione esteri Stefania Craxi per la sua importante relazione.

ci riguarda tutti, perché la libertà delle donne è la libertà di un'intera società, di un'intera Nazione. È importante che questa risoluzione - come diceva prima la presidente Craxi - anche se in ritardo, perché sicuramente la potevamo approvare molto prima, approviamo all'unanimità, così com'è stata approvata in 3a Commissione. È da decenni, ormai, che in Iran donne e uomini lottano con determinazione per ripristinare le condizioni di libertà di democrazia, per il rispetto dei diritti umani. Sappiamo quali sono le torture e anche la dura repressione delle autorità iraniane.

Si contano migliaia di casi, tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che però non hanno soffocato il sentimento di resistenza delle donne e dei giovani per difendere la libertà di ognuno di loro. *(Applausi)*. Come ricordava prima il presidente Craxi, il 13 settembre 2022 quella giovane iraniana di origini curde Mahsa Amini è stata arrestata a Teheran dalla cosiddetta polizia morale della Repubblica islamica e poi - come sappiamo da testimoni oculari - quella polizia morale l'avrebbe picchiata fino a condurla

C'è stata però una grande rivoluzione nel mondo, tante sono state le proteste e finalmente si sono accesi anche i fari mediatici su quello che sta succedendo in Iran, perché quel popolo non va dimenticato in nessun momento; va sostenuto con grande forza, soprattutto dai Paesi occidentali dove noi donne abbiamo la libertà

senza preoccuparci di condizionamenti e di pregiudizi. Appoggiare quindi le proteste del popolo iraniano contro il fondamentalismo è il progetto più grande per chi vuole difendere i diritti delle donne in tutto il mondo. Il giorno in cui le donne iraniane e i giovani che sono accanto a loro in modo particolare distruggeranno il fondamentalismo, la libertà e l'uguaglianza faranno un balzo in avanti in tutto il mondo. mondo. Quelle donne sono scese in campo non solo per la loro libertà, ma anche per liberare un popolo, una Nazione. Per questo dobbiamo essere al loro fianco e sostenerle in ogni momento.

perché vogliono avere anche pieno e libero accesso a Internet e alle piattaforme per la messaggistica istantanea, per comunicare col mondo. Per questo sono importanti i *social media* e tutti coloro che possono accendere questo faro, faro, che è una speranza per quelle donne. *(Applausi)*. Non facciamole sentire mai da sole. Allo stesso modo, dobbiamo chiedere alle autorità iraniane di rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone detenute che sono state arrestate unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel quadro delle attuali proteste. di condannare la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente le libertà e i diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne, nonché le violazioni dei loro diritti politici, sociali, economici e culturali. collaborare con gli organismi della comunità internazionale che hanno avviato missioni conoscitive, per fare piena luce sulle violenze perpetrate in Iran, e proseguire l'intensa azione diplomatica, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e le minoranze presenti nel Paese. a vigilare attivamente sulle operazioni di esportazione di materiali di armamento e munizioni che riguardino anche Paesi limitrofi all'Iran o con i quali esso commerci abitualmente, per scongiurare il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, di aziende italiane nel sostegno all'azione repressiva in atto nel Paese asiatico; asiatico; a sostenere, in accordo con la *policy* dell'Unione europea, le sanzioni in materia di diritti umani in Iran già emesse ed eventuali nuove misure che saranno emanate. Per tutte queste ragioni, non solo sosteniamo le donne, i giovani e tutti coloro che stanno manifestando per la libertà in Iran e, purtroppo, in tanti altri Paesi nel mondo, ma soprattutto chiediamo al Governo un impegno davvero forte - e so che questo impegno ci

Presidente, tramite lei vorrei ringraziare la senatrice Craxi per la relazione che ha introdotto questa discussione e la 3a Commissione per il lavoro che ha fatto e che oggi stiamo approfondendo e discutendo in quest'Aula. vorrei usare una parola che però è difficile usare dovendo parlare di Iran, ma vorrei esprimere la soddisfazione per il fatto che oggi l'Assemblea voti questa mozione - mi auguro unanimemente anche perché credo che sia utile dal punto di vista degli impegni che chiediamo al Governo nello stesso Consiglio europeo dei prossimi giorni, in cui si discuterà nuovamente dell'Iran e delle reazioni che l'Europa deve avere.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel ricevere le credenziali del nuovo ambasciatore dell'Iran nel nostro Paese, ha espresso non solo ovviamente la sua condanna delle violenze,

Non si ricorda nella storia della Repubblica e nella storia della sua Presidenza un'altra occasione in cui il Presidente abbia usato un'espressione di questo tipo. Credo che siano una modalità e un significato assolutamente straordinari, di cui tener conto anche per misurare la distanza tra il comportamento diplomatico che ha tenuto il nostro Paese, a partire dal Presidente della Repubblica, e invece gli argomenti arroganti che il nuovo ambasciatore continua ad esprimere in tutte le occasioni pubbliche. Sempre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a parlare di Iran il 6 marzo, definendo la Repubblica islamica dell'Iran come «un regime che soffoca i propri figli». È un'espressione utilizzata per indicare non solo la repressione che c'era, ma anche una cosa letterale: il lungo elenco delle violazioni dei diritti umani che si sono esercitate in questi mesi in quel Paese è stato ulteriormente alimentato dall'avvelenamento delle ragazze e delle bambine nelle scuole. Credo che nessuno di noi riesca a immaginare un Paese, un Governo o un regime che decidono di provare ad avvelenare le proprie studentesse nelle scuole, nei *campus*, esattamente per punirle della loro volontà di libertà e di autodeterminazione. Forse dovremmo ragionare con più approfondimento su questi elementi, perché pensiamo a quello che, rispetto all'istruzione delle ragazze, sta succedendo nel vicino Afghanistan, e quindi di come in realtà il tema del diritto all'istruzione delle donne sia uno dei tanti elementi che riguardano la condizione, la repressione e la discriminazione nei confronti delle donne in tutto il mondo. Credo che dobbiamo ricordarcene, quando parliamo di rifugiati e di necessità di vie sicure, perché proprio da quei Paesi vengono molti dei rifugiati che non riusciamo a salvare. Non vorrei continuare a percorrere ciò che ci riconsegna quotidianamente la cronaca, anche se penso sia un dovere civile per ognuno e ognuna di noi tenere la lampadina accesa su quello che succede in quel Paese, anche con semplicità, seguendolo sui *social*, continuando a ritwittare, dando il segno che li stiamo vedendo e che non è semplicemente altro da noi. Credo che vada sempre sottolineato quali sono le vittime della repressione che è in corso in Iran: le donne, le giovani donne, esempio esplicito, insieme alla repressione dei giovani, della negazione del futuro; le arti, in tutte le loro forme, dal ballare al cantare, all'esprimersi con le immagini, all'informazione. Se ci pensate, in un Paese di lunga e straordinaria cultura, come quella persiana, è la negazione delle loro radici. Dobbiamo anche guardare con attenzione alle molte minoranze etniche, che sono molteplici in quel grande Paese e oggetto di una repressione peggiore di quella che non si svolga nella capitale. Anche qui, vi è la negazione di una cultura inclusiva. Credo che ci sia, dentro questa repressione delle minoranze, un'ulteriore spina anche per noi: noi Occidente, che abbiamo applaudito i curdi quando combattevano l'Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), abbiamo guardato con rispetto il coraggio delle donne curde che si battevano in quella guerra. Possiamo dirci che un minuto dopo le abbiamo dimenticate, sotto i bombardamenti turchi nella zona del Rojava, ma anche quando sono in prima fila in Iran a battersi per la loro libertà? Eppure, l'inclusione e il rispetto sono un punto fondamentale per poter dire anche noi che applichiamo fino in fondo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. dell'uomo. Abbiamo bisogno anche di ragionare sul fatto che distrarci da quanto avviene in Iran potrebbe essere un problema anche più serio di quello che ci immaginiamo. Noi ci mobilitiamo per l'Iran innanzitutto per democrazia e libertà, per rispetto della vita umana, per la stima e il riconoscimento del coraggio delle giovani e dei giovani iraniani che, con i loro corpi disarmati, con i loro canti, con le loro danze e togliendosi il velo, sfidano un regime che risponde con le armi, con la morte e con la carcerazione. Ci sono anche altre ragioni per guardare con grande attenzione a quello che succede in quel Paese. Credo che una prima valutazione che dovremmo fare è sulle caratteristiche di una rivoluzione della politica che le giovani iraniane hanno determinato: le modalità, la trasversalità e il coinvolgimento che non davamo per certi e che non conosciamo fino in fondo nella loro capacità di essere un grande movimento orizzontale, senza *leader*. Avremmo tutti detto, qualche mese fa, che proprio quella condizione orizzontale senza *leader* sarebbe stata la loro rapida sconfitta; eppure, oggi sembra essere la loro forza. forza. Proviamo poi a interrogarci su quella pervicace convinzione che esprimono e dimostrano della loro disponibilità a morire, a mettere a disposizione la loro vita, convinti che potranno davvero rovesciare quel regime e determinare un'altra storia. Riusciamo noi a immaginare un sacrificio di questo tipo? Siamo capaci di vederlo negli occhi di quei ragazzi e di quelle ragazze della diaspora che incontriamo nelle nostre strade, che sono coraggiosi e determinati e ci dicono con un'assoluta tranquillità e uno straordinario rigore la loro disponibilità e la disponibilità dei loro concittadini, giovani uomini e donne che stanno in Iran, a sacrificare la vita per non dover continuare a vivere in quel regime? Basterebbe indubbiamente questo per vederli, riconoscerli e fare tutto ciò che ci chiedono, che chiedono al Parlamento e al Governo, per aiutarli nella loro lotta. C'è ancora un'altra ragione: non dobbiamo distrarci vedendo l'Iran come un luogo isolato, ma dobbiamo guardarlo nella geopolitica che si sta determinando. Da quel settembre in cui Mahsa Amini ha perso la vita per colpa delle guardie islamiche, l'Iran ha attuato un accordo con l'Arabia Saudita, che si dice patrocinato dalla Cina. l'Iran continua a fornire droni alla Federazione Russa, che vengono utilizzati contro l'Ucraina. Sono state recentemente svolte esercitazioni tra l'Iran, la Russia e la Cina. Sono tutti regimi - non c'è dubbio - che ignorano la democrazia e negano la libertà dei cittadini, ma certamente non sottovalutiamo questo cambiamento politico. Per concludere, vorrei sottolineare due delle questioni che proponiamo al Governo. vigilare sull'esportazione di materiali di armamento e munizioni. Non facciamo questa esortazione a caso, perché vogliamo scongiurare il coinvolgimento diretto o indiretto di aziende italiane, perché ancora dobbiamo fare luce su come le munizioni della Cheddite siano finite nelle piazze dell'Iran. La seconda è dichiarare i *pasdaran* organizzazione terroristica, non solo per sostenere il Parlamento europeo, non solo per guardare negli occhi le ragazze e i ragazzi della diaspora, che ce lo chiedono in tutte le occasioni in cui si mobilitano, ma per un'altra straordinaria ragione. I guardiani della rivoluzione, i *pasdaran*, sono un grande potere economico in Iran e dichiararli organizzazione terroristica non è solo chiamarli con il loro nome, è anche, invece di far soffrire un popolo, dargli le risposte di possibile libertà. *(Applausi)*. «Donna, vita, libertà», tradotto concretamente nelle nostre azioni.

Signor Presidente, tengo anch'io a ringraziare la relatrice, il presidente Craxi, e tutti gli onorevoli senatori. Riguardo agli interventi che mi hanno preceduto, posso assicurare che il Governo italiano ha agito e sta agendo con la più grande fermezza, per condannare un

il Senato approvi la risoluzione in esame è un ulteriore atto di vicinanza importantissimo, direi essenziale, per un popolo che costantemente viene

Governo, la proposta di risoluzione che oggi portiamo alla vostra attenzione rappresenta un atto di amore e di solidarietà verso un popolo che, con tutta la forza di cui è capace, sta cercando la strada della libertà, della dignità e dell'autodeterminazione. un popolo, quello iraniano, che con il suo sacrificio sta conquistando la strada della democrazia e del rispetto dei diritti umani. Ancora abbiamo viva la memoria dell'uccisione della ventiduenne iraniana di origine curde, Mahsa Zina Amini, arrestata a Teheran dalla polizia morale per la presunta inosservanza della legge sull'obbligo del velo. Mahsa muore sotto il tallone di ferro di una dittatura teocratica, che negli anni ha procurato migliaia di vittime. 120.000 sono i casi, tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che pure non hanno soffocato quel sentimento di resistenza che non è mai mancato nel movimento delle donne e del popolo iraniano. Mahsa Amini, spinta in un furgone dalla polizia, picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara, a Teheran, dove poco dopo è entrata, è deceduta il 16 settembre 2022, in un vicino ospedale, mentre si trovava in stato di fermo. terribile la sua storia, che parla di soprusi e violenze quotidiani contro le donne e gli uomini d'Iran, un popolo in ostaggio che chiede al mondo di schierarsi. Questo è il loro urlo. Questa risoluzione intende appunto rappresentare la voce del nostro Paese; intende chiedere al Governo di esercitare la necessaria pressione a livello internazionale e nelle sedi multilaterali affinché si ponga fine alla spirale di violenza e oppressione in Iran, soprattutto ai danni della popolazione femminile e verso le opposizioni e le minoranze presenti nel Paese. Questo provvedimento chiede all'Esecutivo di scongiurare l'esecuzione delle sentenze di condanna a morte comminate dalla magistratura nei confronti dei manifestanti arrestati in questi mesi di proteste e di rilasciare i prigionieri arrestati nel corso delle manifestazioni. Infine, si chiede che venga fatta luce sulla violazione dei diritti fondamentali e sulle violenze che ancora oggi vengono perpetrate ai danni della popolazione civile. L'Iran è diventato una potenza locale anche grazie agli armamenti che continuano a nutrire l'arsenale del Governo di Teheran e, se vogliamo sostenere la popolazione locale nella propria legittima opera di resistenza alla dittatura, è necessario vigilare - di concerto con gli altri Paesi europei - sulle operazioni di esportazione delle armi, anche al fine di scongiurare un coinvolgimento, anche indiretto, del nostro Paese e delle sue aziende nelle operazioni di repressione dell'opposizione interna. L'Italia, i Paesi democratici, il mondo intero non possono essere complici dei crimini dello Stato iraniano. Non possiamo più volgere lo sguardo altrove; non possiamo più essere indifferenti. Il Governo iraniano dev'essere sanzionato per la violazione puntuale e costante dei diritti umani. Schierarsi vuol dire far esprimere il nostro Parlamento e il nostro Governo a sostegno della legittima aspirazione delle donne e del popolo iraniani alla libertà, alla giustizia sociale, alla democrazia. con uno *slogan* che ha attraversato le piazze del Paese e che evoca un sogno di emancipazione per tutto il popolo iraniano: donna, vita, libertà. Voglio infine ricordare che noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, a gennaio scorso, abbiamo avviato il patrocinio politico per salvare i giovani iraniani in carcere. È anche e soprattutto per questo che esprimo con estrema convinzione il nostro sostegno alla risoluzione da noi proposta.

il territorio dell'Iran, nel corso dei millenni, ha ospitato civiltà che hanno costituito un esempio per tutte le altre popolazioni umane del pianeta e sta vivendo una fase di terribile regressione a cui stiamo tutti assistendo, grazie ai *media* che in questo periodo storico ci consentono di farlo. che proprio in Iran, per la prima volta nella storia, un movimento di protesta contro un regime sia innescato da donne che chiedono il rispetto dei loro diritti. In un Paese dove persiste l'obbligo del velo, la disoccupazione femminile è il doppio di quella maschile e per lunghi anni la polizia morale ha controllato ossessivamente i comportamenti femminili, siamo davanti a un fatto di grande importanza storica: da un lato, questa è l'ennesima riprova che i sentimenti di libertà e di uguaglianza sono insopprimibili per l'essere umano; dall'altro, questa è la conferma di quanto forti siano questi sentimenti nelle donne, non più disposte a vedere la loro vita e il loro corpo come strumenti piegati al fondamentalismo politico e religioso. Il regime ha reagito, in questo caso, come tutti quei regimi che si sono trovati davanti a eventi inattesi e vissuti come peccato di lesa maestà: ma chi sono queste ragazze e anche questi ragazzi che si permettono di mettere in discussione l'ordine costituito? Dove trovano la forza? Perché non si spaventano? Perché gli atti di disobbedienza crescono di ordine e di numero? Ne è scaturita una repressione di inaudita violenza, con carcerazioni, torture e condanne a morte, davanti alla quale

convocando al Quirinale l'ambasciatore iraniano in Italia. Bene facciamo noi oggi a votare questa risoluzione, che condanna in modo netto gli eventi e soprattutto dà un mandato molto chiaro al Governo per attivare tutti i canali allo scopo di mettere fine alle violenze e per scongiurare il rischio di un coinvolgimento anche indiretto di aziende italiane nell'azione repressiva in atto. Il nostro compito non si esaurisce però di certo qui. Come Senato, siamo chiamati a tenere alta l'attenzione di tutto il nostro Paese su una mobilitazione che progressivamente sta coinvolgendo tutta la società iraniana. Lo dobbiamo fare per difendere i diritti universali in Iran e in senso lato nel mondo, ma anche per far sentire la nostra vicinanza a quelle ragazze e a quelle donne che, con il loro coraggio, stanno mandando un messaggio straordinario anche alle donne dell'Afghanistan e a tutte quelle che vivono, in tanti Paesi, in una condizione di oppressione e di privazione dei più elementari diritti. Annuncio pertanto il voto favorevole del nostro Gruppo alla risoluzione.

Tanti sono i condizionali usati e tanti i fatti riportati, come ovviamente sulla stampa. La prudenza in questi casi è d'obbligo, considerate le diverse fonti d'informazione, che vanno valutate. Per capirci, se oggi chi si trova all'estero dovesse leggere alcuni titoloni e articoli di alcuni giornali italiani contro il Governo italiano, potrebbe pensare che sia responsabile del naufragio di Cutro; ma sappiamo benissimo che non è così. Va valutata anche l'evoluzione che nel frattempo si è avuta in Iran su diversi aspetti su cui si focalizza la risoluzione, che è la stessa dal dicembre 2022. Questa è una premessa per evidenziare che le conoscenze dirette di quanto sta accadendo sono diverse e spesso contrastanti; è fondamentale quindi capirne la reale portata. Come sempre accade, sappiamo che a una notizia ne è sempre contrapposta un'altra. Molti dei fatti che vengono narrati stanno anche nella dinamica tra Governo e opposizione iraniana. Siamo certi di una cosa: l'Iran - o, meglio, la Persia - che conoscevamo non è più tale, ha subito un'evoluzione dopo l'avvento della Repubblica islamica. È però un fatto che ci siano stati importanti moti di piazza per cambiare e arrivare a maggiore libertà. La risoluzione è quindi prudente, ma anche concreta negli impegni del Governo italiano, impegni che certamente condividiamo. Stiamo attenti a non usare troppo la parola "democrazia". Troppi sono stati ormai i tentativi di imporre la democrazia da parte dell'Occidente e altrettanti sono gli insuccessi che sono seguiti a quei tentativi, in varie parti del mondo. Il mondo diviso in buoni e cattivi, come lo conoscevamo prima, non c'è più e noi, come Italia, dobbiamo fare in modo che certe alleanze tra Paesi e certe saldature di interessi non avvengano in chiave antioccidentale. Bisogna certamente lasciare che la coscienza del popolo iraniano cresca, bisogna fare in modo che la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero sia garantita, proprio per far crescere questa coscienza. Stiamo attenti a non fare gli errori già commessi dall'Occidente in Afghanistan o in Libia, tanto per citare gli esempi più eclatanti e di cui subiamo le conseguenze, anche con le ondate migratorie. Vanno certamente evidenziate la recente pace diplomatica siglata tra Iran e Arabia Saudita e la riapertura delle rispettive sedi diplomatiche, proprio a indicare nuovi equilibri mondiali: a mediare questo accordo è stata la Cina, che ormai si impone anche come superpotenza diplomatica. L'ostilità tra Iran e Arabia Saudita ha per lungo tempo provocato danni in larga parte del Medio Oriente. La Regione mediorientale ha visto coinvolti in queste ostilità l'Iraq, il Libano, la Siria e lo Yemen. La ripresa dei rapporti è un'ottima notizia e ha ridotto l'isolamento in cui era finito per mesi il Governo iraniano. Condividiamo anche l'impegno sul controllo del percorso delle armi. L'Italia, che è uno dei principali produttori di armi al mondo, deve avere su questo punto un ruolo preciso: ne conosce i mercati internazionali, è in grado di valutare eventuali triangolazioni e cessioni nel mercato nero; nero; deve evitare quindi che le proprie armi finiscano in mani sbagliate o, peggio, di essere complice di eventuali traffici. L'invito è dunque a usare le fonti certe e la diplomazia per riportare l'Italia al centro di una seria e concreta azione diplomatica. Ci riconosciamo certamente

Il fatto che a metà febbraio il Governo iraniano abbia concesso un'amnistia a oltre 20.000 manifestanti e abbia graziato in totale più di 80.000 iraniani coinvolti nelle proteste indica un'ulteriore presa di coscienza di Teheran. Certamente bisogna lavorare ancora per porre fine a ogni eventuale forma di repressione, per fermare ogni tipo di violenza e di danni alle donne, ai pacifici manifestanti e alle minoranze etniche e religiose. Bisogna quindi fare in modo che che vi sia un accesso libero e non condizionato dei cittadini iraniani sia all'informazione, sia a *Internet*, sia alle piattaforme per la messaggistica istantanea. Certamente la diplomazia può sempre avere un ruolo per scongiurare il rischio che venga dato corso all'esecuzione delle sentenze di condanna a morte comminate nei confronti di alcuni manifestanti arrestati, un ruolo da esercitare soprattutto attraverso le decisioni e le risoluzioni nei consessi internazionali. In questo senso, è fondamentale la collaborazione con gli organismi della comunità internazionale, alcuni dei quali hanno già avviato missioni conoscitive per fare piena luce sulle violenze commesse in questi mesi ai danni dei manifestanti in Iran. Ciò che tuttavia potrà portare a maggiori risultati - lo di proseguire un'intensa azione diplomatica. L'obiettivo è convincere il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e per tutte le minoranze presenti nel Paese.

Signora Presidente, qualcuno un giorno mi ha detto che i diritti civili sono il canarino dei minatori.

se gli animaletti cominciavano a soffocare e a morire, significava che l'ambiente stava diventando tossico; era l'allarme per i minatori che le prossime vittime sarebbero stati loro. I diritti delle donne sono il canarino per eccellenza. Ovunque nel mondo i primi diritti a essere violati e conculcati sono immancabilmente quelli delle donne. La spia della trasformazione di uno Stato in regime totalitario e illiberale è data dalle leggi che colpiscono la libertà delle donne, i loro spazi, la loro salute riproduttiva e la loro partecipazione alla vita politica, sociale ed economica. La loro violazione è così diffusa e pervicace che in un certo senso abbiamo accettato il fatto che in molte parti del mondo si pratichi, in gradazioni diverse, un'*apartheid* di genere: alcune leggi valgono per gli uomini, altre valgono per le donne. Tutti i luoghi sono in genere consentiti agli uomini, solo alcuni alle donne. In Iran non va diversamente. L'*apartheid* di genere non è però un'esclusiva dell'Iran, come la polizia morale non è una sua istituzione esclusiva. come spesso accade, l'ennesima violenza compiuta da parte di quest'ultima - la polizia morale - è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. Il massacro di Mahsa Amini, avvenuto per un *hijab*, un velo, a loro dire indossato male, e il goffo tentativo del Governo di far passare la sua barbara morte per un incidente provocato un'ondata d'indignazione che si è trasformata in imponenti manifestazioni pacifiche che, a partire dal 16 settembre scorso, ancora non si fermano. La risposta del regime, però, è stata ancora una volta brutale. Da sei mesi le donne iraniane guidano le proteste, chiedendo libertà, diritti e democrazia. Le parole d'ordine sono: "Donna, vita, libertà". Un trinomio di origine curda, a quanto si sa, e assolutamente adeguato. Le donne danno la vita e la vita, senza libertà, non ha senso, si spegne. Nelle rivolte generate dalla violenza, reazione delle autorità iraniane, sono state uccise oltre 750 manifestanti e 30.000 persone sono state arrestate. Ora, se è vero che ogni cambiamento non può che provenire dal popolo iraniano stesso e dalla sua resistenza, è pur vero che la comunità internazionale non può non fare tutto quanto in suo potere per sostenere le donne iraniane e gli uomini che sono al loro fianco. I gruppi di resistenza iraniana che tutti, in quest'Aula, abbiamo qualche volta incontrato ci chiedono di non voltarci dall'altra parte. Siamo ben consapevoli dei delicati equilibri internazionali in gioco, ma la *realpolitik* deve trovare un punto d'incontro con la naturale propensione umana di stare al fianco di chi combatte per i propri diritti e per la propria libertà, anche al rischio della propria vita. Dall'ultimo rapporto del Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran, è emerso che le migliaia di persone arrestate nelle carceri iraniane a seguito delle proteste, tra le quali anche diversi cittadini europei ed occidentali, subiscono condizioni di detenzione inumane. Sono soggetti a torture e sono stati condannati addirittura alla pena di morte, dopo procedimenti giudiziari sommari, privi delle più elementari garanzie processuali.

Spesso sono ragazze e ragazzi giovanissimi, di appena diciannove o vent'anni, di cui tuttora ignoriamo la sorte. I movimenti di resistenza iraniani chiedono il riconoscimento dei diritti individuali e sociali ricompresi nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di pensiero, di parola e di stampa, la libertà di organizzarsi politicamente, il divieto di torture e l'abolizione della pena di morte. Il MoVimento 5 Stelle appoggia queste richieste e sostiene con forza le aspirazioni di autodeterminazione del popolo iraniano, che vuole vivere in un Paese libero, stabile, inclusivo e democratico, che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali, a partire da quelli delle donne. Ci uniamo alle richieste di questo Parlamento, di condannare con fermezza la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili, attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente libertà e diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne, nonché le violazioni dei loro diritti politici economici, sociali e culturali. Chiediamo pertanto al Governo italiano di non essere timido e di intensificare l'azione diplomatica di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani delle proprie cittadine e dei propri cittadini, inclusi quelli delle minoranze presenti All'inizio di questo mio intervento dicevo che i diritti civili e quelli umani sono il canarino dei minatori. Quando il canarino muore, vuol dire che l'ambiente è tossico e che rischi di morire anche tu. Per questo, quando ovunque nel mondo, anche nel nostro Paese, vengono messi in discussione i diritti acquisiti delle donne, nessuno può scrollare le spalle e dire che è roba da donne e che ci pensino loro. Per questo, quando ovunque nel mondo, anche nel nostro Paese, si negano i diritti e le tutele delle persone LGBT, nessuno può dire: non mi riguarda, io non sono gay, non sono mica lesbica. Quando il canarino dei diritti muore, vuol dire che l'ambiente è tossico e che la prossima vittima potesti essere tu.

rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla cessazione dell'azione repressiva delle manifestazioni pacifiche conseguenti la morte di Mahsa Amini. Permettetemi di ringraziare innanzitutto la presidente Craxi e tutti i membri della Commissione per il loro contributo, che ha portato alla stesura di questo importante documento. Consentitemi anche di esprimere vicinanza all'amica europarlamentare Cinzia Bonfrisco, entrata nella *black list* dell'Iran, perché, vorrei ricordarlo, è stata la prima firmataria di una lettera inviata a novembre all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di di sicurezza Borrell, la quale ha portato alla risoluzione, con l'esclusione dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sulle condizioni delle donne. Cinzia Bonfrisco da allora è entrata quindi nel mirino del regime. regime, secondo Amnesty International, dall'inizio delle manifestazioni di ottobre dello scorso anno ha portato alla morte di oltre 500 persone, di cui una settantina sono bambini. È un regime che non si ferma nel condannare a morte donne incinte o che consente alle proprie forze di sicurezza di prenderle a calci nella pancia facendo perdere loro il bambino. Essere nel mirino di un regime come quello iraniano fa paura,

Purtroppo non è l'unica barbarie. Sempre secondo Amnesty International, le forze di sicurezza e di *intelligence* iraniane hanno commesso orribili atti di tortura, tra cui percosse, fustigazioni, stupri, scosse elettriche ai testicoli contro bambini manifestanti di appena dodici anni. A questi vanno aggiunti i fenomeni di avvelenamento di migliaia di studentesse avvenuti nell'ultimo mese, oggetto di un'interrogazione depositata dal Gruppo Lega ed oggetto anche di una risoluzione votata dal Parlamento europeo la scorsa settimana. L'ONU ha formulato accuse nei confronti delle autorità in Iran che e, secondo il rapporto del relatore ed osservatore dei diritti umani, sono basate su accertamenti di gravi violazioni della libertà con violenze accertate e omicidi compiuti nei confronti dei manifestanti che ultimamente stanno cercando di dimostrare il dissenso al regime imposto. Sono state identificate come le peggiori violazioni dei diritti degli ultimi quarant'anni. L'Iran sta vivendo da molti anni una condizione dove la *sharia* genera oppressione, oscurantismo, degrado sociale ed economico, ma più di ogni altra cosa il Paese è una terrificante prigione per le donne che vivono segregate da un regime religioso teocratico e fondamentalista. però non è sempre stato così: possiamo trovare fotografie che ritraggono ragazze iraniane sorridenti, truccate e con i capelli al vento, donne libere. Queste immagini non rappresentano soltanto le condizioni delle donne, ma il livello di civiltà e libertà di un popolo.

diciotto anni l'età per il matrimonio, fu limitata la poligamia e fu introdotto il diritto delle donne al divorzio, attraverso la riforma del codice di famiglia. Con la rivoluzione iraniana del 1979 però e la trasformazione dell'Iran in una Repubblica islamica la cui Costituzione si ispira alla legge coranica e alla *sharia*, le donne sono state quelle che ne hanno pagato maggiormente le conseguenze. fu immediatamente segnato, a partire dalla reintroduzione dell'obbligo del velo e dall'abbassamento dell'età per il matrimonio a nove anni, con l'abolizione appunto del codice di famiglia. Mi chiedo quale credo o quale dio possano autorizzare un uomo ad obbligare una bambina di nove anni a sposarlo e quale uomo possa trovare naturale abusare di una bambina. Questo non è essere uomini. Questo non è credere in qualcosa o in qualcuno, il termine giusto è pedofilia e, come tale, dev'essere duramente combattuta. *(Applausi)*. Le proteste a settembre dello scorso anno, che hanno visto l'uccisione di Mahsa Amini, hanno evidenziato il malessere delle donne iraniane e non solo. Contrariamente alle altre proteste avvenute in passato, oggi in Iran assistiamo a un fenomeno che si è diffuso a macchia di leopardo in tutto il Paese, coinvolgendo ampie fette della popolazione, a prescindere dall'età, dal genere e dall'appartenenza sociale. Molto significative sono le parole contenute in un messaggio rivolto al popolo iraniano dal filosofo sloveno Slavoj Zyzek nel commentare le rivolte iraniane: gli uomini che partecipano alle manifestazioni «Donna, vita e libertà» sanno bene che la lotta per i diritti delle donne è anche la lotta per la propria libertà. L'oppressione delle donne non è un caso speciale, è il momento in cui l'oppressione che permea l'intera società è più visibile. Questo a me pare il punto centrale: laddove le donne non hanno cittadinanza, i diritti di ogni essere umano sono in pericolo. I diritti delle donne sono alla base dei diritti universali e non ci sono diritti universali dove non c'è la completa separazione della religione dallo Stato: la libertà di religione o di credo è un importante diritto umano, è una questione di coscienza; quando però la religione è parte integrante dello Stato o della legge non si tratta più di credo personale, ma di potere e controllo sulla collettività. La difesa della laicità è una sfida importante per i progetti islamisti che aumentano in Europa, come le corti della *sharia,* il *burqa* o la segregazione di genere nelle università britanniche. Ebbene, proprio partendo dal messaggio del filosofo vorrei fare una riflessione su quello che accade anche in Italia: penso al caso Saman, ai tanti matrimoni forzati e alle donne con il *burqa* sempre più presenti nelle nostre città. Abbiamo visto un'involuzione proprio in questo senso: mentre fino a qualche tempo addietro in Italia le donne con il *burqa* erano pochissime, oggi sono molte. signora Presidente, rubo le parole di Oriana Fallaci: «C'è molto sole sui Paesi dell'Islam, un sole bianco, violento, che acceca. Ma le donne musulmane non lo vedono mai: i loro occhi sono abituati all'ombra come gli occhi delle talpe. Dal buio del ventre materno esse passano al buio della casa paterna, da questa al buio della casa coniugale, da questa al buio della tomba».

ed aggiungo che aiutiamo anche quelle che vivono in Italia a far sì che proprio in casa nostra non vengano nuovamente avvolte dal buio. *(Applausi)*.

È il modo in cui possiamo testimoniare la vicinanza più alta di coloro che rappresentano il popolo italiano, al Senato come alla Camera,

manifestazione che poteva diventare davvero virale nel suo passaggio su Internet. Non a caso, le piattaforme per messaggistica di Internet più utilizzate dai più giovani sono state il primo obiettivo del regime. Già le aveva vietate nel 2009, quelle più conosciute e più diffuse (penso a Facebook e Twitter), ma lo ha subito fatto nei giorni successivi a fine settembre, provando a cercare di arginare un moto di popolo che invece non si è fermato, perché il passaparola funziona ancora, al di là delle tecnologie, ed è stato impetuoso,

dalla zona del Kurdistan iraniano. Poi si è diffuso qualcosa di imprevedibile, perché si è saldata la protesta dei più giovani e delle donne, che inizialmente bruciavano il velo e si tagliavano

le richieste profonde di cambiamento nei confronti di una società oppressiva, nella direzione delle libertà, soprattutto dei diritti fondamentali delle donne, dei più giovani e delle giovani generazioni, con le proteste di alcuni strati popolari, certamente in difficoltà per le pesanti sanzioni occidentali, soprattutto durante il regime di Ahmadinejad. Queste proteste diverse si sono saldate, ma non hanno ancora trovato il favore di alcuni strati: penso ad alcuni settori lavorativi, ad esempio quello del gas e del petrolio, in cui la morsa del potere e del regime è ancora molto forte. La reazione del regime è stata devastante: quella di chi ha paura di perdere tutto davanti a una morsa che mette insieme le migliori energie del Paese, ma anche appunto strati popolari profondamente scontenti della loro situazione economica e che si sentono abbandonati ed emarginati. È una miscela esplosiva, i cui esiti possono essere i più nefasti. Il regime, oltre a intervenire in maniera

agenzie delle Nazioni Unite, non si è fermato e ha raggiunto il culmine a dicembre e a gennaio con esecuzioni capitali di giovani e anche l'uccisione di minori e donne, di ragazzine (penso a mia figlia che ha sedici anni), per il solo fatto di aggiustarsi il velo in maniera diversa, sono state uccise dalla repressione.

che avevano l'unica colpa di voler chiedere maggiori libertà e manifestare per i diritti civili. Da questo punto di vista, serve una reazione forte di tutto il mondo occidentale. Le Nazioni Unite hanno avviato le loro indagini su un elemento davvero inquietante, com'è stato già ricordato: l'intossicazione di migliaia di ragazzi e di studentesse, su cui il regime ha abbozzato all'inizio. Poi, davanti a una manifestazione ampia che raccoglieva sicuramente il consenso di tante parti e anche di quelle preoccupate dalle manifestazioni, ha dato una prima risposta, ma è stata evasiva e non sufficiente. Ora, che cosa fare? Questo è il punto e anche diversi analisti si interrogano su quello che sta succedendo e su quello che può provocare anche qualche mossa sbagliata da parte dell'Occidente. Ricordavo ieri, in dichiarazione di voto, come

l'accordo raggiunto con i responsabili della sicurezza iraniana e saudita: un tentativo di riunificare. In passato vedevamo le foto dei Presidenti americani fra Sadat e Begin (quello era il turno di Carter). Poi abbiamo visto,

il popolo iraniano. Sono tutti ragionamenti che vanno fatti, anche dal Governo italiano e in ambito europeo, su come vogliamo agire, utilizzando gli strumenti della diplomazia internazionale, per evitare che l'Iran venga sempre più attirato dall'egemonia cinese. Hanno già partecipato a esercitazioni militari congiunte, fanno parte - perché gli è stato richiesto - dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e da questo punto di vista non è facile intervenire, però l'Europa ha il vantaggio di poter insistere, appunto, sull'accordo sul nucleare per arrivare ad allentare le sanzioni sul popolo iraniano e allo stesso tempo, però, perché noi siamo diversi da questo punto di vista, esercitare il *soft power*. Da questo punto di vista, possiamo offrire un modello diverso rispetto alla Cina, che è quello - con una battuta - del *business* senza diritti. Noi abbiamo un'arma fondamentale nella politica estera italiana, che certamente è quella della cooperazione; ci sono la politica commerciale, l'azione politico-militare, la partecipazione nelle operazioni di *peace-keeping*, ma anche la lotta, la tutela e la difesa dei diritti umani e dei principi fondamentali. In quello siamo diversi e dobbiamo dimostrare in tutte le sedi

Ha ragione la collega Camusso quando dice che non a caso vengono colpite le giovani generazioni e le donne, che rappresentano una speranza per il futuro. Non a caso vengono colpite vengono colpite le diverse forme d'arte, il libero pensiero, la possibilità che qualcuno la possa pensare in maniera diversa, perché quella è la prima crepa per i regimi. La forza dei regimi è la possibilità di contare sull'omertà delle persone. delle persone. Coloro che stanno manifestando, mettendo a rischio la propria vita, devono quindi sapere che in Italia, come in Europa e nei Paesi occidentali, ci sono altre persone che non fanno calcoli, non applicano il realismo politico che spesso viene applicato nelle relazioni internazionali di politica estera, ma sanno che questa volta si gioca una partita per la libertà e i principi; quelle stesse libertà e principi che sono scolpiti nelle nostre Costituzioni e che abbiamo il dovere di difendere, a fianco di quelle donne e di quegli uomini che con coraggio manifestano per la libertà. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare ed esprimere, anche da parte di Fratelli d'Italia, un vivissimo apprezzamento alla presidente Craxi, a tutti i colleghi della Commissione esteri e ai colleghi che hanno parlato in questo momento, per aver assunto l'iniziativa di una risoluzione che è importante per una serie di motivi.

Abbiamo citato il caso di Masha Amini, ma migliaia e migliaia di donne, di dimostranti e di persone sono state incarcerate, impiccate e torturate in Iran negli ultimi cinque-sei

nel khomeinismo di uno Stato che è teocratico, fondamentalista sciita, e che può essere benissimo definito islamico terrorista, come definivamo l'ISIS di matrice sunnita. Uno Stato sciita terrorista, contro il suo popolo e contro i popoli vicini, che ha però la prerogativa di essere un grande Paese fornitore di *business*, di petrolio e di affari a troppa gente che ci va con grande leggerezza, magari perdendoli anche gli affari, è uno Stato che solleva illusioni straordinarie. Consentitemi di dire che anche oggi ne ho sentita qualcuna, cioè che ci sia una riformabilità del regime khomeinista, del *velāyat-e faqih*, del potere dei giureconsulti, dell'identificazione che tutto quello che avviene è la legge di Dio e chi fa qualcosa, anche una contravvenzione stradale, è un apostata, un *mohareb*, una persona da torturare, da impiccare, e lo decidono i giureconsulti.

Khomeyni, Khamenei, Rafsanjani, Montazeri, Khatami, Rouhani e ne potrei citare altri. Tra questi ci sono i più riformisti che il Paese abbia prodotto, che hanno continuato ad impiccare a più non posso. Rouhani, il grande riformista, era quello che uccideva e impiccava più persone, ogni giorno, di ognuno dei suoi predecessori *(Applausi)* e abbiamo fatto affari, mandato delegazioni e sollecitato l'Unione europea.

Per questo motivo, ascoltando le dichiarazioni di voto, ho il piacere di constatare oggi, non certo per i pochissimi accenni che ho fatto anche ieri su questo tema, l'importanza di una maggior coesione, ampiezza e base parlamentare per i grandi temi di politica estera. *(Applausi)*. Questo è uno dei grandi temi di politica estera. È un tema che riguarda l'Ucraina, perché l'Iran è combattente sul terreno in Donbass, con sue milizie, reclutate in Siria, Afghanistan e Yemen. Con i suoi droni, le sue armi e i suoi missili ammazza gli ucraini direttamente, non per interposta persona. Queste milizie sono comandate dal corpo dei *pasdaran*, dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Non facciamo finta di non sapere tutto questo. Lo sappiamo benissimo, non l'abbiamo letto solo sui giornali, ma in molti casi l'abbiamo ascoltato di persona.

a Villepinte, quattro anni fa, penso che eravamo stati oggetto di un attentato mostruoso. Un diplomatico, accreditato all'ambasciata iraniana a Vienna, Assadollah Assadi, processato perché colto con un esplosivo ad altissimo potenziale, che stava portando all'interno di quell'aula, dove c'erano tante persone, perlomeno con una trentina di amministratori locali, di personalità, di giornalisti, di parlamentari italiani.

è stato condannato a vent'anni di reclusione, il massimo della pena in Belgio, ma si cerca naturalmente di scambiarlo e l'Iran cattura poveri innocenti, che acchiappa in giro per il mondo, che transitano dai Paesi vicini, per tenerli in carcere e scambiarli con Assadollah Assadi. Era è una persona che, in due anni, aveva fatto centottanta viaggi in Europa, era capo di una rete terrorista iraniana ed era un diplomatico iraniano. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui si pone un problema serio. Vogliamo continuare a fingere che tutto questo non esista? Vogliamo lasciare scorrazzare queste bande iraniane in giro per l'Europa e anche in Italia? Vogliamo lasciare che continuino a uccidere personalità politiche, dissidenti politici, persone *(Applausi)*, uomini, donne, ragazzi, che siano davanti ai loro carnefici?

della società iraniana: una società giovane, splendida, di gente magnifica, di grandi intellettuali, di persone di enorme coraggio. Dobbiamo parlare con loro; ci sono grandi organizzazioni: quella guidata dalla signora Rajavi è una di queste; è quella che raccoglie più sostegno all'interno del Paese probabilmente, ma ce ne sono anche altre; sono democratici con carte vere, credenziali serie. Se andiamo a visitare i loro luoghi - anche in Albania sono rappresentati -

30.000 martiri dei *mujaheddin*, del popolo soprattutto, anche di altre etnie, non soltanto politiche, ma etnico-culturali del Paese. I *mujaheddin* del popolo hanno perso 30.000 persone impiccate da una commissione che rispondeva a una *fatwa* dell'*ayatollah* Khomeini. E da chi era guidata la commissione della morte? Penso che molti lo sappiano: dall'attuale presidente della Repubblica islamica Raisi. Su questo Iran non dobbiamo illuderci; ci dev'essere un segnale forte da parte della comunità internazionale. Mi ha fatto piacere sentire la senatrice Camusso

Le forze della sicurezza iraniana controllano più della metà dell'economia del Paese. Per questi motivi, perché quanto fatto con questa risoluzione è un passo importante, ho l'onore di dichiarare il voto favorevole di Fratelli d'Italia, nell'auspicio che sia un voto unanime di tutta l'Assemblea.

il documento in esame prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia.

In base alla disciplina istitutiva in esame, la Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari e con la garanzia di almeno un componente per ogni Gruppo. Sono inoltre stabilite le disposizioni sulla costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione e sull'adozione del regolamento interno e si specifica che le sedute della stessa sono pubbliche, eccettuati i casi in cui la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta. Per l'adempimento delle proprie funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato e può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra, occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti (il documento demanda al regolamento interno la definizione del numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione). I compiti di accertamento della Commissione sono individuati analiticamente dall'articolo 3. Si ricorda, in via di sintesi, che essi riguardano: l'entità dello sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione; la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, alla sussistenza di differenze tra i sessi, tra le fasce di età, tra le aree territoriali e i settori lavorativi, nonché con particolare riguardo agli interventi di assistenza prestati alle vittime e alle loro famiglie;

della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; *c*) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti; l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro; l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla sicurezza sul lavoro; l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche; l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro per i lavoratori e le loro famiglie, per la produttività delle imprese, per il Servizio sanitario nazionale e per il sistema economico; l'incidenza della formazione permanente, l'efficacia dell'istruzione scolastica e universitaria e universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione in Italia rispetto agli altri Paesi; gli eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il documento disciplina, poi, i poteri e i limiti della Commissione, i quali, in conformità al principio costituzionale sulle Commissioni parlamentari di inchiesta, sono definiti con riferimento a quelli per le autorità giudiziarie; la modalità di acquisizione di atti e documenti e il regime di segretezza degli stessi; l'obbligo generale del segreto sugli atti di inchiesta per i commissari, il personale addetto e gli altri collaboratori o gli altri soggetti che partecipano o vengono a conoscenza di tali atti. PRESIDENTE.Grazie, senatore Magni. Nonostante l'emozione della prima volta, abbiamo apprezzato la sua relazione.

Presidente, intervengo solo per dire che sono davvero molto contento che tutta l'Aula abbia votato favore degli articoli che istituiscono questa Commissione e che, presumibilmente, farà lo stesso quando si tratterà di esprimere il voto finale.

di quanto siano intervenute una serie di profonde modifiche strutturali che hanno significativamente, in qualche caso addirittura clamorosamente, cambiato l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione del lavoro, rendendola molto diversa da quella che conoscevamo in passato. Intorno a una diversa organizzazione del lavoro, si è evidentemente definita e strutturata anche una società particolarmente diversa, ma questi mutamenti hanno generato anche una enorme, in qualche caso drammatica, frammentazione che certamente non aiuta e anzi spesso mette le lavoratrici e i lavoratori in una condizione di maggiore difficoltà e anche una materia come quella relativa alla sicurezza delle condizioni di lavoro in qualche modo ha profondamente a che fare con questi elementi di frammentazione.

gentili colleghi, gentile Sottosegretario, credo di capire bene l'emozione con cui il senatore Magni ha voluto aprire la discussione e credo che non fosse solo legata al luogo nel quale presentava

questo è stato il primo disegno di legge che ho voluto presentare come senatore e l'ho voluto fare anche simbolicamente, rispetto alla mia precedente esperienza di amministratore locale come assessore al lavoro del Comune di Bologna. Oggi siamo contenti di affrontare una votazione che, al di là delle appartenenze ai Gruppi politici, riconosce l'utilità dell'istituzione di una Commissione di inchiesta. Vorrei che la parola giusta, che purtroppo è risuonata anche in quest'Aula per vicende diverse estere, risuonasse nella sua crudezza anche rispetto all'argomento trattato e la parola è "guerra". Presidente, ogni giorno muoiono tre persone in Italia sul luogo di lavoro e non ci sono solo i morti, ci sono anche gli infortuni sul lavoro che sono oltre 600.000 l'anno; stiamo parlando di oltre 2.000 infortuni al giorno; giorno; sono i numeri di una guerra. Questi sono i numeri ufficiali che l'INAIL ci dà ogni anno in occasione del 22 ottobre, la Giornata nazionale per riflettere sul tema, ma non è detto che questi siano i numeri che davvero certificano la realtà, perché purtroppo sappiamo che esistono tanti casi di infortuni sui luoghi del lavoro che non vengono neanche certificati come tali. Il voto di oggi significa che per noi tutti lavorare non può

questi numeri sono il segno di un tradimento del sogno dei nostri Padri costituenti che volevano porre il lavoro a fondamento della nostra vita democratica e della nostra comunità. Riaffermare i diritti sui luoghi di lavoro, a partire dalla vita e dalla salute, è un generatore di valore per la società. Con questa Commissione non solo abbiamo il dovere di continuare a lavorare sul monitoraggio, sull'informazione e sulla prevenzione, ma a mio avviso abbiamo anche il dovere culturale di evitare l'assuefazione evitare l'assuefazione sui numeri dei morti e degli infortuni sul lavoro. Evitiamo l'assuefazione rispetto alla contabilità. Morire sul lavoro non è mai una fatalità: evitiamo anche l'utilizzo di termini che non descrivono la verità. È una sconfitta per tutti, è una ferita sociale che lacera il Paese, ma non è una ferita sociale che lacera le nostre coscienze; se fosse così anche noi, in quest'Aula, a volte non saremmo complici di alcune delle cause che determinano gli infortuni sul lavoro. Tutti noi, infatti, sappiamo benissimo che dove c'è lavoro precario il rischio di infortunio sul lavoro è più alto e che tutte le volte che non contrastiamo la precarizzazione del lavoro, aumentiamo l'incidenza dei rischi di infortunio e di decesso;

Noi dovremmo essere consapevoli che il costo della sicurezza non può essere un elemento di competizione economica. Quando determiniamo il tema del minor costo delle gare al massimo ribasso, dobbiamo essere consapevoli che le prime voci di taglio che vengono fatte sono quelle sul costo del lavoro, sulla sicurezza e sulla formazione. Quando non riusciamo a contrastare il fenomeno delle cooperative di comodo o delle cooperative spurie, che sono molto attive nei settori della logistica e dell'agricoltura, non riusciamo a determinare le condizioni per le quali ci può essere sicurezza nei luoghi di lavoro. Dobbiamo sapere che quando non riusciamo a contrastare i contratti collettivi di comodo, cioè quelli non fatti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

cerchiamo di far luce sul perché non eravamo pronti a valutare la sicurezza nei luoghi di lavoro a causa della pandemia. Evitiamo che lo stesso problema si possa ripetere, come ci dicono le organizzazioni internazionali e le strategie che richiedono investimenti nelle infrastrutture per la resilienza. Ce lo fanno capire temi sui quali non vorrei che noi, per distrazione, superata l'emergenza della stretta fase pandemica, non cogliessimo il lavoro che c'è da fare sulla prevenzione e sulla formazione. Questo non lo si può fare per parti separate: lo devono fare tutti i partiti politici insieme e lo devono fare le istituzioni, l'ispettorato del lavoro, le autorità locali, le amministrazioni locali, le organizzazioni sindacali. Si tratta di una guerra da combattere tutti insieme come sistema Paese. Paese. Vorrei che questo fosse un ambito dell'attività di questa Commissione di inchiesta: non solo assumere tutte le informazioni che possono essere utili al Parlamento per legiferare e per rendere effettive le misure di controllo, ma riuscire anche a fare un lavoro di sensibilizzazione per non essere noi indifferenti rispetto ai numeri sui decessi rispetto ai numeri sui decessi e sugli infortuni, rispetto ai numeri di una guerra silenziosa che il nostro Paese purtroppo ogni giorno si trova ad affrontare. Ripeto, ci sono tre morti al giorno dichiarati e più di 2.000 infortuni sui luoghi

Di questa proposta credo sia doveroso apprezzare il fatto che non verrà trattato soltanto il tema degli infortuni sul lavoro o della sicurezza, come nelle precedenti Commissioni infortuni; temi ancora centrali, naturalmente, ma lo spettro di indagine della nuova Commissione sarà molto più ampio. Oggi dobbiamo riconoscere che il testo ampliato dal lavoro della 10a Commissione ha messo a fuoco nuove e ulteriori tematiche da approfondire, come ad esempio la differenza tra sessi nel mondo del lavoro, argomento che porta con sé altri temi estremamente attuali come la parità di retribuzione o il diritto ad avere congedi parentali. La 10a Commissione ha inoltre aggiunto un punto importante di cui occuparsi, che riguarda la digitalizzazione e l'impatto delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza del lavoro. Voglio infine sottolineare la questione della formazione, il collegamento di questa col percorso di studi, il raffronto tra il livello di formazione italiano e quello estero. Questo nuovo perimetro di lavoro definito per la Commissione di inchiesta è uno scenario che oggi abbiamo il dovere di sostenere, perché permetterà al Parlamento di poter avere una lente di ingrandimento su tutti gli aspetti attuali, sui quali è giusto accendere una luce neutrale e terza. Tutto ciò permetterà al legislatore di comprendere le criticità e offrire spunti per migliorare le condizioni di lavoro di tutti i cittadini italiani. L'obiettivo, quindi, dovrà essere quello di analizzare, studiare e mettere a disposizione, con il consenso più vasto possibile, una serie di puntualizzazioni sulla legislazione vigente. Forza Italia ha da sempre posto la questione lavoro come tema centrale di tutti i programmi di Governo e delle iniziative politiche intraprese, sia quando siamo stati all'opposizione, sia quando siamo Nel rispetto dei valori, degli ideali e di quella tradizione che da sempre accompagna le nostre battaglie, oggi siamo qui a sostenere la costituzione di questa Commissione, che riteniamo utile e indispensabile in avvio di questa XIX legislatura. Il nostro impegno non mancherà, soprattutto sui temi della semplificazione, che ritengo debbano tornare a essere centrali nelle politiche sul lavoro e incidere positivamente nella vita di ogni lavoratore di questo Paese. Per queste ragioni, con estrema convinzione annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza-Berlusconi Presidente. Signor Presidente, dico in partenza che il MoVimento 5 Stelle appoggia pienamente l'istituzione di questa Commissione di inchiesta. Presidente, noi in questo momento abbiamo delle emergenze gravi da risolvere in questo Paese

Il lavoro povero: oggi abbiamo 4,5 milioni di lavoratori poveri, persone che, nonostante lavorino, non riescono ad uscire dalla condizione di povertà. Eppure, quando parliamo di salario minimo, ancora ci viene detto che è impossibile inserire il salario minimo legale e che basta invece rafforzare la contrattazione collettiva. Abbiamo l'emergenza lavoro precario: oggi i lavoratori precari sono oltre 3 milioni e moltissimi di questi sono giovani.

Questo chiaramente spinge moltissimi giovani ad andare via: sono oltre 120.000 i giovani che ogni anno lasciano il nostro Paese per non fare più ritorno e spesso sono giovani anche altamente formati. Abbiamo certamente l'emergenza dei servizi al lavoro, che purtroppo in questo Paese non esistono: le cosiddette politiche attive del lavoro. Negli anni abbiamo investito appena lo 0,03 per cento del PIL; pensiamo che la Germania investe dieci volte tanto. Vorrei ricordare che le Regioni che hanno la competenza sui servizi al lavoro non sono nemmeno riuscite a spendere il miliardo di euro che avevamo stanziato in legge di bilancio 2020 per assumere i lavoratori nei centri dell'impiego *(Applausi)*, che sono i luoghi deputati ai servizi al lavoro. Certamente tra le emergenze da affrontare per il lavoro ci sono le condizioni dei lavoratori e i turni massacranti. Penso, ad esempio, ai lavoratori del comparto sanitario: li abbiamo costretti a lavorare in condizioni estreme, li abbiamo chiamati eroi, eppure ancora non sono partiti i censimenti per stabilizzare i tanti lavoratori precari *(Applausi)*, nonostante abbiamo fatto delle leggi che permettono alle Regioni di stabilizzare chi abbia maturato diciotto mesi di lavoro durante la pandemia. la pandemia. Questo lavoro così precario, così sottopagato, così massacrante, con turni che non sono tollerabili, è evidente che causi anche dei problemi di sicurezza. Qui parliamo di una vera e propria mattanza, Presidente, come ricordavano i miei colleghi: più di mille morti all'anno sul lavoro, quasi tre morti al giorno. Le chiamiamo "morti bianche", ma di candido non hanno assolutamente nulla. Spesso sono giovani; è capitato che a morire fossero anche giovani durante l'apprendistato o il tirocinio, spesso sono madri o padri che escono per andare al lavoro e non fanno più ritorno nelle proprie famiglie. Questa Commissione di inchiesta deve avere - a nostro avviso - tre obiettivi principali. Il primo è quello della formazione: a questo Paese, purtroppo, manca la costruzione di una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro, che secondo noi deve partire dalla scuola. Per questo abbiamo depositato un disegno di legge che istituisce l'insegnamento della sicurezza sul lavoro già nel percorso scolastico. Il secondo obiettivo fondamentale è quello della prevenzione, Presidente, anche in questo campo l'arma più potente che abbiamo e che come Stato possiamo mettere in campo è certamente quella della prevenzione. ci sentiamo dire che investire in prevenzione è troppo costoso, ma non si tiene conto che quegli investimenti a lungo termine significano certamente risparmio di spesa in termini di invalidità. Il terzo obiettivo fondamentale è quello della conoscenza e dell'informazione: conoscenza di quali sono i comportamenti corretti da seguire; conoscenza e informazione anche su quegli incidenti che si chiamano *near miss*, ovvero quasi incidenti, che spesso non vengono neppure registrati, eppure sono proprio l'indicatore di una condizione lavorativa in sicurezza, oppure non in sicurezza, o in sicurezza apparente. Presidente, riteniamo che bisogna anche fare un altro passo, con l'istituzione di una vera e propria procura nazionale del lavoro *(Applausi)*. Ci stiamo provando dalla scorsa legislatura: purtroppo non abbiamo mai avuto i numeri per approvare questa proposta di legge, perché anche su questo siamo stati sempre isolati Eppure, avere una procura nazionale sul lavoro, con dei magistrati che seguono quegli infortuni, renderebbe molto più rapide tutte le indagini successive, che oggi invece richiedono moltissimo tempo. Signor Presidente, oggi abbiamo un'idea di lavoro che andrebbe totalmente stravolta, ma credo che un po' i nostri giovani stiano andando in quella direzione. Oggi i giovani parlano di

guadagnare per vivere, andrebbero totalmente riviste: il lavoro deve diventare un valore aggiunto, uno strumento che permetta a ciascuna persona di realizzare il proprio progetto di vita, il proprio sogno. Questo è quello a cui dovremmo mirare. Ricordiamolo anche quando diciamo ai nostri giovani tutto sommato dovrebbero accontentarsi di qualsiasi lavoro venga loro offerto. Lo abbiamo fatto tutti, signor Presidente, ma tutti poi abbiamo avuto e dobbiamo avere l'ambizione di realizzare, anche attraverso il lavoro, il nostro sogno, il nostro progetto di vita. Potremo fare le leggi più belle del mondo ma, se non capiamo che la società non può guardare solo alla produttività, non avremo mai davvero un futuro migliore.

Signor Presidente, illustrissimi colleghe e colleghi, la tematica della sicurezza sul lavoro ritorna in Assemblea, finalmente, perché purtroppo le statistiche sono terribili. Circa 6.300 persone muoiono ogni giorno nel mondo a causa di incidenti sul lavoro o malattie professionali. Condivido quanto detto dalla collega Castellone, del Gruppo MoVimento 5 Stelle, che l'emergenza non sono i *rave party*. Ebbene, cara collega, non lo sono più grazie alla legge voluta dal Governo.

con l'obiettivo di arrivare a zero morti sul lavoro, come diceva il sottosegretario Durigon. Già nella scorsa legislatura, alla Camera dei deputati, in Commissione lavoro, si erano incardinate alcune proposte di legge, di cui ero stata relatrice, ma dopo audizioni varie, a causa del Covid-19 e di altre urgenze, non si è potuti arrivare a una conclusione. Istituire una Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza è importante. Si tratta di temi importanti, che voglio analizzare in dettaglio. Prima di tutto si parla delle condizioni di lavoro, nei vari ambienti e settori, per verificare i diversi contratti che vengono applicati, perché sappiamo benissimo che esistono contratti pirata o contratti inadeguati al luogo o alla mansione che una persona viene chiamata a svolgere. Già è stato fatto in agricoltura con la Commissione di inchiesta sul caporalato, nella scorsa legislatura, ma quello è solo un ambito, purtroppo, di contratti irregolari e di sfruttamento. Basta aprire un quotidiano locale: indagini della Guardia di finanza vengono fatte ogni giorno, e a loro va il nostro elogio per il loro operato. Purtroppo, scoprono situazioni irregolari o di lavoro nero in diversi ambiti e settori. Per non parlare delle gare d'appalto, dove si parla di massimo ribasso, il cui primo taglio arriva proprio dal costo del personale o, infine, delle cooperative spurie, che applicano condizioni contrattuali illecite e sono le stesse cooperative regolari - possiamo chiamarle così ci chiedono di arrivare direttamente a una situazione per vagliare e migliorare il loro operato. È importante analizzare nella Commissione anche la sicurezza sul lavoro a 360 gradi, con un ampio e incisivo intervento di semplificazione e aggiornamento del testo unico sulla sicurezza sul lavoro e del sistema assicurativo, anche sotto il profilo della vigilanza.

per adempiere a infinita burocrazia, togliendo in tal modo tempo alle reali verifiche che devono essere fatte e sottraendo risorse necessarie alla formazione, che è una tematica importante su cui bisogna investire. Infatti, come si suol dire anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro, prevenire è meglio che curare. Concludo, Presidente, ritenendo necessaria e fondamentale questa Commissione, per la quale, per il Gruppo Lega, annuncio il voto favorevole. Tuttavia, riteniamo altrettanto necessario e fondamentale arrivare alla conclusione dei lavori della Commissione non solo con una relazione, ma anche con un atto concreto e condiviso che porti a cambiamenti veritieri per giungere a condizioni regolari per tutti, con la conciliazione di vita, lavoro e famiglia, prospettive di contratto innovativo di un mercato del lavoro che cambia ed è flessibile, ma soprattutto - come dicevamo - con l'obiettivo morti zero.

colleghe e colleghi, tramite lei, Presidente, vorrei ringraziare il relatore e la 10ª Commissione per il lavoro fatto. Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico, vorrei anche sottolineare che mi pare si possa dire che questo sarà un voto unanime dell'intera Assemblea; il che rende quella di istituire una Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro una scelta impegnativa per il Parlamento; una scelta impegnativa per il Parlamento; una scelta che deve partire dal fatto che vi sono nel nostro Paese alcuni milioni di lavoratori e di lavoratrici che vivono in una condizione di precarietà, perché fanno il *part time* involontario, perché hanno contratti brevissimi, magari solo di alcuni giorni. Bisogna sapere che, quando si ha un contratto a termine che dura solo alcuni giorni, per esempio, la formazione obbligatoria non viene fatta, perché non c'è il tempo materiale per farla. Bisogna sapere che, se ci si abitua all'idea di contratti che continuano a essere reiterati per brevissimo periodo, ciò significa che l'investimento sulla formazione e sulla sicurezza non c'è. Non si può avere l'idea che una formazione compiuta per affrontare i temi della sicurezza possa avvenire nella logica del temporaneo, breve, del meno costoso possibile. Sto parlando di lavoro legale, neanche di tutto quel mondo, che invece esiste, indubbiamente, di lavoro informale o di lavoro nero. Il problema è che più si destruttura il lavoro e i suoi diritti, più si riduce la sicurezza; più si riduce la qualità del lavoro più, in realtà, si introduce l'idea di un sistema di produttivo, di un sistema di servizi che non è in grado di dare certezze ai lavoratori. Questo anche perché, per esempio, quando si fa un codice degli appalti che prevede il subappalto a gogò come se nulla fosse, si introducono grandi elementi di ricattabilità dei singoli lavoratori che, di fronte alla necessità, rinunciano anche a pretendere condizioni sicure di lavoro. Il lavoro, quindi, non è insicuro soltanto perché possono presentarsi imprevisti e imprevedibilità. Il lavoro spesso è insicuro perché non lo si conosce o non lo si affronta e perché non si investe in termini di prevenzione e condizioni positive. Nel documento che ci apprestiamo ad approvare per insediare la Commissione ci sono molti impegni, che sono indicati nell'articolo 3 - come ci ricordava il relatore hanno l'idea, che io credo sia fondamentale, che nessuno dei temi riguardanti le condizioni di lavoro può essere isolato rispetto agli altri. C'è una trasversalità, c'è una relazione tra la sicurezza e il tipo di contratto che hai, c'è una relazione tra la sicurezza e il tipo di formazione che hai. Dobbiamo anche cominciare a ragionare sul fatto che c'è una relazione tra la sicurezza e le trasformazioni tecnologiche che sono in atto in termini di cambiamento dei sistemi produttivi, ma forse anche in termini di opportunità. Vorrei soffermarmi per un momento su uno dei temi che abbiamo affidato a questa Commissione, di cui si parla in genere solo in occasione della Giornata internazionale: il lavoro minorile. Noi diamo in qualche modo per scontato che nel nostro Paese questo tema non ci sia. Non è vero. Lo diciamo perché in realtà non abbiamo alcuna rilevazione statistica che ci permetta di dire se esiste o non esiste il lavoro minorile nel nostro Paese. Nel 2021 i consulenti del lavoro indicavano in 2,4 milioni i lavoratori che avevano cominciato a lavorare prima dei sedici anni. Nel 2019 l'Ispettorato del lavoro rileva, durante le sue ispezioni, 243 casi di illiceità dal punto di vista dell'età; di nuovo, ne rileva altri 127 del 2020 e poi non abbiamo altri dati. Possiamo sempre pensare che sia un fenomeno minoritario. La verità è che, per esempio, una delle attività a cui potrebbe dedicarsi la Commissione di indagine è iniziare a rilevare statisticamente questo fenomeno e a vedere come possiamo intervenire affinché non ci sia quella che io considero un'onta sull'immagine del nostro Paese e sulla sua scelta rispetto al lavoro. Come dicevano già altre colleghe e colleghi, si lavora per vivere e non si vive per lavorare. Nessun lavoro può chiedere alle persone di perdere la salute o, ancora peggio, la vita. Eppure, c'è una strage che si ripete anno su anno e che troppo spesso si risolve in qualche minuto di ricordo o in qualche ora di cordoglio, ma non diventa mai un tema centrale dell'iniziativa. Il dato del 2022 (l'ultimo dato disponibile) ci dice che gli infortuni sono stati 697.773 e che sono aumentati del 25,7 per cento rispetto al 2021; che gli incidenti mortali sono stati 1.090, più di tre al giorno. So che qualcuno ha commentato dicendo che siamo di fronte a una lieve differenza rispetto al 2021 e al 2020. Purtroppo quella differenza è data dal fatto che la pandemia da Covid è stata anche un acceleratore delle morti sul lavoro. quota consistente (oltre mille morti ogni anno) di incidenti che si ripetono negli stessi settori e con le stesse caratteristiche, che si ripetono da circa sessanta anni. dobbiamo dedicare e contemporaneamente dobbiamo sapere che crescono, e spesso non le riconosciamo, le malattie che derivano dal lavoro, quelle che chiamiamo malattie professionali, così come crescono le patologie da lavoro correlato. correlato. Questa Commissione, allora, non è solo un luogo per riepilogare le cose che già conosciamo o quelle che magari non conosciamo (per esempio che nel 2021 gli infortuni femminili sono cresciuti del 42,9 Aumentano in generale, per uomini e donne, gli infortuni *in itinere*; forse vuol dire che si corre troppo, ci si deve troppo spostare per rincorrere i lavori e viene meno la sicurezza.

Allora cosa possiamo fare per affrontare il fatto che esistono delle dinamiche di infortunio che continuano a ripetersi? Credo che non possiamo continuare a dire che l'unico strumento è quello della formazione. La formazione è sicuramente uno strumento essenziale, ma non è l'unico. Dobbiamo esplorare quel mondo nuovo, di cui spesso diamo di per sé un giudizio positivo: il mondo delle tecnologie, dell'innovazione, del digitale. È un mondo che ci offre grandi contraddizioni. Quello dei *rider* non è un lavoro sicuro, anzi, abbiamo purtroppo la testimonianza di come sia molto pericoloso. Ci sono invece altre situazioni in cui la tecnologia sui cicli produttivi ha determinato la riduzione delle condizioni di sicurezza, delle tecnologie è un mondo vasto. Per esempio, potremmo ragionare sul fatto che, se non si entrasse in una cisterna quando i sensori indicano la presenza di gas, forse non si ripeterebbero degli infortuni che c'erano prima?

basta che il lavoratore sappia e questo di per sé impedisce che si generino infortuni. Non basta che il lavoratore o la lavoratrice sappiano. Non possiamo cioè non ragionare sulla gravità

Forse abbiamo bisogno di rimettere energie, fantasia, proposte e di cogliere l'insieme di quelle trasversalità che indagare sulla sicurezza sul lavoro, ma soprattutto abbiamo bisogno di prevenire e di determinare condizioni sicure. Credo che in fondo possiamo dirci che questo è uno dei migliori compiti che può essere affidato a un'Aula parlamentare. È una delle migliori espressioni di potestà legislativa alla quale possiamo ambire

Signor Presidente, colleghi, quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è da sempre un tema di grande centralità nel nostro Paese e si condivide pienamente la necessità di trovare soluzioni in grado di ridurre il numero di infortuni e di vittime, purtroppo ancora molto alto. La proposta in esame tratta - come si è già detto - molte tematiche complesse e solo apparentemente slegate tra loro, in quanto gli incidenti sul lavoro sono spesso correlati alla legalità o, meglio, all'illegalità del lavoro. Troppo spesso ci si occupa delle cosiddette morti bianche solo in occasione degli eventi di cronaca più eclatanti, dimenticando che ogni giorno decine di lavoratori vengono coinvolte in incidenti sul lavoro, spesso non correttamente identificati. Responsabilità della politica è quindi occuparsi del tema con continuità e programmazione su tutto il territorio nazionale, con riferimento a tutti comparti, consapevoli che gli infortuni pesano in modo rilevante dal punto di vista economico e gravano sul sistema sanitario, previdenziale, assicurativo, amministrativo e giudiziario. La sicurezza è da considerarsi, pertanto, un investimento in positivo e non meramente un costo e questo passaggio necessita di un cambio culturale importante. Le cause alla base degli infortuni sul lavoro sono molteplici. Sicuramente rilevanti sono le cause organizzative (legate a un processo di ammodernamento tecnologico, di macchine e di attrezzature), la scarsa prevenzione, la disattenzione e la superficialità spesso legata a scarsa informazione e formazione dei lavoratori e, in particolare, l'illegalità, perché gli infortuni aumentano proprio laddove ci sono meno controlli e comunque in realtà imprenditoriali dove prolifera il lavoro nero o sommerso. L'orientamento maggiormente utilizzato sino ad oggi, ovvero il solo approccio repressivo, non basta. Vanno sviluppate e incentivate tutte le politiche di carattere preventivo. Per fare ciò serve davvero un cambio culturale. Investire in sicurezza non significa necessariamente spendere in sicurezza: investire in sicurezza ripaga ampiamente a livello aziendale, ma soprattutto a livello sociale (spesa sanitaria, previdenziale, assicurativa). Sul tema della consapevolezza e della cultura della sicurezza, pur riconoscendo che l'Italia è dotata di un quadro normativo certamente avanzato, potrebbe essere opportuno riflettere sulla realizzazione di una campagna mediatica che metta al centro del suo messaggio l'importanza della prevenzione. È necessario incentivare l'ammodernamento tecnologico, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, potenziando e sfruttando al meglio anche le iniziative e le agevolazioni promosse dall'INAIL. riconoscere, valorizzare e incentivare gli sforzi delle aziende virtuose che operano nel rispetto delle regole e che investono in sicurezza. Occorre migliorare l'informazione. È indispensabile avere un sistema informativo moderno e aggiornato, conoscere non solo gli infortuni indennizzati dall'INAIL, ma anche i rischi a cui i lavoratori sono esposti, comprendendo anche quelli in condizione di fragilità, rapporti di lavoro variegati, instabili, orari e turni, che vanno ad aggiungersi ai normali rischi lavorativi; tanto più oggi alla luce dei profondi cambiamenti del mondo del lavoro che hanno spostato il baricentro del luogo stesso, definito ormai da una pluralità di possibili luoghi di lavoro. Occorre far dialogare tutti i dati disponibili; banche dati dell'INAIL, del Ministero della salute, dell'Istat,

strumento culturale di prevenzione perché coinvolgere e responsabilizzare lo stesso lavoratore rispetto ai pericoli è fondamentale. La sua consapevolezza e la sua preparazione sono la prima neutralizzazione del rischio, dove non si può operare l'eliminazione totale alla fonte. una formazione di qualità. Taluni operatori della formazione spesso offrono alle aziende servizi formali, non effettivamente formativi, e questo svuota il significato dell'obbligo formativo a tutto svantaggio delle imprese sane, che invece sostengono importanti costi per una formazione permanente, Grazie a tutti accompagnato da politiche sanzionatorie eccessivamente onerose, va rivisto, mentre va potenziata la vigilanza là dove vi sia il sospetto di coinvolgimento di lavori invisibili, in nero o comunque rapporti non regolari. È opportuno che gli interventi ispettivi prendano in considerazione soprattutto queste realtà imprenditoriali e lavorative al fine di supportare le imprese che intendono mettersi a norma e individuare quelle che operano nell'illegalità. In tale direzione si colloca proprio il piano nazionale per l'emersione del lavoro sommerso, approvato dal Governo a dicembre. La sfida sarà soprattutto quella di rendere superiore per le imprese i benefici dell'operare nella legalità rispetto ai costi connessi all'utilizzo del lavoro irregolare, rendendosi a tal fine necessario un *mix* di procedure di prevenzione e promozione del lavoro regolare accanto a una ridefinizione delle misure di deterrenza. È sempre quindi necessario ricercare il giusto equilibrio tra l'esigenza delle aziende e la tutela circolare dei diritti dei lavoratori. Ciò significa dare dignità e valore a chi lavora, garantendo il rispetto di orari, riposo, formazione e professionalità, senza però dimenticare che la centralità del lavoratore è sul fronte non solo dei diritti, ma anche dei doveri, intesi soprattutto come attenzione e responsabilizzazione, fattori necessari per fronteggiare e prevenire in maniera adeguata il rischio di infortuni gravi. Dall'altra parte, le imprese devono avvertire la presenza di uno Stato che supporta e aiuta perché la sicurezza deve essere patrimonio collettivo. Il dialogo sociale su una materia così delicata è avvertito anche dall'opinione pubblica. Oggi più che mai dobbiamo investire tutti: le istituzioni, ad ogni livello, le organizzazioni sociali di rappresentanza, i corpi intermedi e la stessa società civile. Per tutte queste ragioni, annuncio il parere favorevole del Gruppo Fratelli

Risultano pertanto assorbiti i documenti XXII, nn. 5, 6 e 11.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

Quest'anno il tema è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. Il messaggio è ridurre gli sprechi e assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Stiamo vivendo un allarme mondiale e il fatto che la siccità si stia protraendo da ormai due anni ci induce a riflettere sulle nostre responsabilità e sul nostro modo di abitare la terra e di non considerare che le risorse sono scarse. Occorre mettere in relazione tra loro le risorse, considerandole interdipendenti e facenti parte di un unico grande ecosistema: l'acqua con il suolo, il suolo con le piante, le piante con l'aria e l'aria con il suolo. Ed occorre comprendere che danneggiare una parte significa finire per danneggiare le altre. Come ricordato il 21 aprile scorso nella risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo, il suolo è l'ecosistema più essenziale di tutti.

il suolo è l'ecosistema più essenziale di tutti. Quindi, se manca l'acqua è anche perché trascuriamo i suoli, che potrebbero trattenerla. Perché consumiamo il suolo, alterando il ciclo delle acque, con tutti i danni che ne conseguono? Perché siamo pervicacemente fissati su agricolture intensive, non più ammissibili e perché promuoviamo una dieta alimentare super idroesigente. Occorre, dunque, avviare cambiamenti radicali nel nostro stile di vita e indurre le nostre economie a fare altrettanto. Urbanizzare un prato significa rinunciare a far infiltrare un quantitativo di acqua fino a quattro o cinque volte di meno e questo aggrava gli effetti della siccità. Lo deve sapere l'urbanista e lo deve sapere il sindaco che approva un piano urbanistico con nuove e vecchie urbanizzazioni. Il 50 per cento della pioggia si infiltra solo se incontra superfici a prato o a bosco. Se queste diminuiscono, specie in pianura, è un grave problema. La metà dell'acqua che si infiltra scende giù in falda e l'altra metà rimane nei primi centimetri di suolo. Dobbiamo pensare ad una grande cisterna, che accumula acqua preziosa per restituirla poco alla volta alle piante. Quindi, anche quando non piove, soprattutto quando non piove, tutta l'acqua che rimane in campo è acqua preziosa che non perdiamo. Se, invece cementifichiamo, le poche acque di pioggia scorreranno via velocemente; e se la pioggia sarà intensa e breve, rischiamo pure di fare gravi danni. Un suolo non urbanizzato può trattenere fino a 3,8 milioni di litri di acqua, ovvero 150 TIR di bottiglie di acqua. Quindi, queste sono buone ragioni per parlare, proprio nella Giornata mondiale dell'acqua, dell'azzeramento, ora, del consumo di suolo. La Giornata dell'acqua non serve per invocare la pioggia, ma per capire che la politica deve darsi da fare per avviare i necessari cambiamenti radicali.